Signor Presidente, onorevoli senatori, la manovra di bilancio che vi presento oggi si iscrive in un disegno politico delineato è un anno e da allora perseguito con coerenza e con tenacia. Sedovessi condensare in una sola frase il senso di tale disegno, direi che abbiamo voluto restituire all'azione di governo l'ampiezza di un progetto che partendo dall'oggi guardi lontano nel futuro. Potrebbe sembrare un proposito scontato, ma un esame sereno convince che così non è. Per troppi anni è stato commesso l'errore di affrontare i problemi dell'oggi ipotecando le risorse del domani; per troppo tempo è sembrato che la saggezza e la bravura consistessero, come in un rodeo di cavalli, nel restare in sella rinunciando a darsi una direzione. L'origine dell'immenso debito pubblico dell'Italia è tutta in questo errore di prospettiva. E così pure l'origine della fiacchezza della nostra crescita economica. Per dare un domani all'Italia dobbiamo operare guardando lontano ma senza curarci del nostro domani. La scorsa legislatura si aprì con promesse mirabolanti, ma si concluse con la scomparsa dell'avanzo primario, la risalita del debito, l'incoraggiamento aperto all'evasione fiscale, il sacrificio degli investimenti in infrastrutture a favore della spesa corrente, l'ingresso in una rischiosa procedura di infrazione delle regole europee; una procedura per noi particolarmente pericolosa proprio perché il debito - che per oltre la metà è in mano di investitori esteri ci rende esposti sul mercato internazionale come nessun altro Paese. Le vere anomalie della finanza pubblica italiana, alle quali anche questa manovra cerca di porre riparo, si riducono a due. La prima è il gigantesco debito pubblico, il più alto in Europa e il terzo al mondo in valore assoluto: 1.600 miliardi di euro che ci obbligano a reperire ogni anno circa 70 miliardi per il pagamento dei relativi interessi; 1.200 euro all'anno, in media, in testa ad ogni italiano, compresi i neonati. La gara europea la iniziamo ogni anno con 5 punti di penalizzazione rispetto ad agguerritissimi concorrenti. La seconda anomalia è l'ampiezza dell'evasione fiscale, anch'essa del tutto fuori linea rispetto alla media europea. Il divario ammonta a circa 5-6 punti di Prodotto interno lordo: 75-90 miliardi di euro ogni anno. Che nessuno o quasi ponga questi due semplici fatti, sempre e di nuovo, al centro delle sue analisi e dei suoi giudizi è veramente singolare. Ma i fatti sono ostinati e la loro forza alla fine è irresistibile. Rivendico al Governo Prodi di aver posto la questione del debito e la questione dell'evasione fiscale al centro dell'attenzione; e grazie a questo continuo *memento***,** di aver fatto finalmente crescere la consapevolezza del peso che una politica economica miope ha posto sulle spalle innocenti di chi veniva dopo, quelle dei giovani di oggi e di domani. Come si fa strada la consapevolezza che è il cittadino in regola col fisco a pagare, nel senso letterale, se il suo vicino con l'auto di lusso, la terza o quarta casa e magari la barca di altura dichiara redditi da collaboratore domestico o da vigile urbano. Sappiamo che la pressione fiscale è alta in Italia, anche se non più alta di quella dei Paesi a noi vicini. Ma sono del tutto fuorvianti le campagne di propaganda e disinformazione che tendono a presentare il recupero dell'evasione come un aumento delle imposte. No: semplicemente paga il dovuto chi prima non pagava. E oggi, con un anticipo che solo pochi mesi fa non avrei ritenuto possibile, la manovra finanziaria contiene le prime concrete "restituzioni" ai contribuenti di risorse recuperate all'evasione. Mi è particolarmente gradito sottolineare che in questa operazione di recupero, vitale per l'economia e per l'etica sociale del nostro Paese, il personale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sta dando prova di grande impegno e perizia tecnica. Solo la poca stima di sé che affligge noi italiani ci impedisce di giudicare questi due risultati così come li giudicheremmo se riguardassero un altro Paese: successi spettacolari. Grazie a questi due successi abbiamo potuto intraprendere l'alleggerimento fiscale per i contribuenti in regola nonché riprendere gli investimenti nei trasporti per ferrovia, nelle strade, nella ricerca. Oggi possiamo così presentare una manovra finanziaria molto diversa da quella passata. Per la prima volta da molto tempo conseguiamo una riduzione del disavanzo, senza dover effettuare una manovra correttiva. Presentiamo una manovra di restituzione fiscale, di semplificazione, di investimenti, di riqualificazione della spesa pubblica, di rafforzamento del sistema di protezione sociale. Manteniamo tutte le promesse fatte. Siamo in linea con il programma di legislatura e con le risoluzioni parlamentari sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Il Governo è consapevole della sua responsabilità di decisore ultimo; ma proprio questa consapevolezza sorregge la sua convinzione che le scelte condivise siano anche quelle che portano agli esiti migliori. La manovra di bilancio è frutto di una cooperazione con e tra le principali istituzioni e rappresentanze del Paese. Accoglie il risultato di accordi e intese con il sistema delle autonomie locali, con le parti sociali, con il mondo universitario; di incontri e discussioni con i rappresentanti di numerosissimi settori della nostra vita civile ed economica. Ma la manovra è soprattutto il frutto dello sforzo compiuto dagli italiani; sono essi che hanno fatto uscire il Paese dall'emergenza dei conti, dimostrando di accettare sempre più il basilare principio che tutti debbono assolvere al loro compito di contribuenti. Di questo voglio qui ringraziarli. Prima di illustrare gli specifici interventi della manovra di bilancio, debbo esporre l'argomento generale che li ispira. Esso si riassume così: il ritorno a una crescita economica prolungata e sostenibile è la questione centrale. Tornare a crescere è indispensabile per dare una prospettiva ai giovani, per mantenere o raggiungere livelli di benessere, qualità della vita, sicurezza sociale, tutela dell'ambiente, influenza internazionale, corrispondenti all'ambizione di un Paese industriale avanzato. La spinta per tornare a crescere il Paese deve farla scaturire al proprio interno, deve trarla da un desiderio di eccellenza; non gli verrà da sollecitazioni esterne, né di natura economica né di natura politica. Per il Governo ciò vuol dire, in primo luogo, fare buon uso, miglior uso di quanto abbia saputo fare fin qui, delle risorse che i contribuenti gli conferiscono perché produca beni pubblici e servizi alla collettività. In linguaggio economico si dice che la produttività del settore pubblico deve aumentare strutturalmente. È difficile ma possibile. Lo spazio per crescere c'è. Basterebbe che ci allineassimo alla media europea in termini di aumento della produttività e di partecipazione alle forze di lavoro perché l'economia salisse con una crescita annua del 2,5-3 Si dimezzerebbe in meno di un decennio il peso del debito. La grande ingiustizia arrecata alle nuove generazioni sarebbe sanata. Ecco a che cosa serve la crescita. Ecco perché essa è indispensabile in una prospettiva che guardi al futuro e non all'immediato. Per aiutare l'economia a crescere, il settore pubblico ha un ruolo essenziale da svolgere e nello stesso tempo si trova oggi in una condizione molto difficile: anno dopo anno esso ha accumulato debito e mancato di accrescere il capitale fisico e umano di cui dispone per servire il Paese. Anzi, quel capitale lo ha consumato. Di qui la mancanza di strade, che impedisce la mobilità in intere Regioni; materiale ferroviario obsoleto e insufficiente; infrastrutture carenti, università prive di posti per giovani scienziati; uffici scarsi di tecnici e ingegneri. Per un generale salto di qualità, occorre tempestivamente investire. E per investire non possiamo né indebitarci né chiedere più soldi ai contribuenti: dobbiamo risparmiare, economizzare. Per la prima volta lo Stato presenta il bilancio in una forma che rende comprensibile ai cittadini la destinazione delle risorse che essi gli affidano. La nuova classificazione del bilancio si basa su 34 missioni, corrispondenti alle grandi finalità perseguite, che, a loro volta, si articolano in circa 170 programmi che raffigurano il complesso delle attività svolte. La vecchia classificazione era incentrata su chi gestisce le risorse, sulle amministrazioni. La nuova guarda a che cosa si fa con le risorse, le destinazioni, le funzioni. Il bilancio finalmente parla in lingua italiana, diventa leggibile per tutti. Anche la legge finanziaria diventa più leggibile e snella: per ogni singolo programma rende chiare le variazioni di risorse proposte rispetto a quelle già disponibili; ha dimensioni contenute sia nelle cifre, sia nelle norme: 11 miliardi in luogo di 35; 96 articoli in luogo dei 217 del 2007. Contestualmente al bilancio e alla finanziaria, il Governo presenta un decreto-legge che reca misure di restituzione fiscale e di forte sostegno agli investimenti con effetti sul 2007, ma strettamente legato alla logica complessiva della manovra. Entro la metà di ottobre, poi, il Governo presenterà il primo collegato, recante le misure su lavoro e previdenza che recepiscono gli accordi del 23 luglio 2007. Poiché la copertura di queste misure sta nella legge finanziaria, è irrinunciabile per il Governo che le Camere, utilizzando le risorse dei Regolamenti vigenti, come spesso è stato sottolineato autorevolmente, garantiscano la deliberazione definitiva almeno di questo collegato entro il 31 dicembre 2007. La procedura parlamentare sarà facilitata da una limitazione degli emendamenti proposti dal Governo e dal loro raggruppamento. Se la cornice regolamentare in vigore, con il concorso leale e trasparente della maggioranza e dell'opposizione, riuscirà ad assicurare il rispetto di questi termini temporali senza il ricorso alla fiducia, le istituzioni della democrazia repubblicana avranno raccolto in modo adeguato il monito del Primo Magistrato della Repubblica. La legge finanziaria, anche quando ha le ampie dimensioni dell'anno scorso, incide solo su una parte modesta (pochi punti percentuali) delle risorse che passano per i conti pubblici: è solo il mutamento marginale che si apporta ogni anno alle cifre del bilancio dello Stato centrale. È dunque ben poco giustificata l'attenzione spasmodica che si accentra attorno ad essa ed è anche fuorviante, perché porta a concentrare gli sforzi e il dibattito su aspetti spesso secondari. Distoglie dalla questione fondamentale: come vengono impiegate le risorse a disposizione. È da augurarsi che non sia lontano il giorno in cui il disegno di legge di bilancio, che entra in Parlamento il primo giorno di ottobre, non abbia bisogno di una legge finanziaria che lo modifichi. Quel giorno indicherebbe che la legislazione implicante entrate o spese si è evoluta ordinatamente ed efficacemente nel corso dell'annata parlamentare, sicché la sessione di bilancio possa limitarsi a registrarne le implicazioni contabili, così come immaginavano i Padri costituenti. Ma nessuna famiglia, nessuna impresa, nessuna organizzazione gestirebbero le proprie finanze dando sostanzialmente per intoccabili le scelte compiute fino a quel momento, come se il continuo mutamento dei bisogni, delle preferenze, delle tecnologie delle conoscenze non richiedesse una continua revisione dell'intero bilancio. Si impone ormai una revisione progressiva delle modalità d'impiego dell'intero ammontare delle risorse di bilancio. Il bilancio pubblico è risultato di una stratificazione di leggi, pratiche amministrative, strutture organizzative, rapporti tra amministrazioni, società e organi di Governo (centrale e locale), impegni con sindacati, imprese, rappresentanze di categorie. È per molti versi un dato acquisito, arduo da modificare. È per questo che non si può credere ai colpi di magia, alle soluzioni facili; per ottenere risultati in termini finanziari e di qualità dei servizi ci vuole tempo. Occorre saperlo e dirlo con chiarezza: chi propone la colla a presa rapida, ricette immediate e miracolose, se è in buona fede sta ingannando se stesso e, comunque, inganna il suo prossimo: la prova l'abbiamo fatta molto di recente. Con questa manovra di bilancio il riequilibrio dei conti prosegue: il *deficit* si riduce dal 2,4 per cento del PIL nel 2007 al 2,2 per cento il debito pubblico scende dal 105 al 103,5 per cento. Si arresta la crescita della spesa primaria rispetto al prodotto; si ferma la pressione fiscale. Per la prima volta dopo molti anni, la proposta del Governo non ha bisogno di reperire nuove risorse per destinarle al rispetto dei conti e degli impegni europei. I mezzi ricavati dal recupero di imposte evase e dalla riduzione di spese permettono una prima riduzione del carico fiscale, il sostegno di coloro il cui reddito è tanto basso da non comportare obblighi di imposta (i cosiddetti incapienti), l'investimento in capitale materiale e immateriale. Sono coperte le spese che nel DPEF del giugno scorso erano state indicate come dovute, anche se non ancora contabilizzate perché non recepite della legislazione vigente. Il contenimento della spesa pubblica è un obiettivo costante di tanti Governi. Che sia difficile da conseguire lo sa perfettamente chiunque vi si sia accinto. È invece facile predicarlo ogni giorno dalle tribune, alimentando l'illusione e rendendo così il compito ancora più arduo. Che limitare la spesa sia possibile lo dimostra un fatto incontestabile: vi sono Regioni, Comuni, ospedali, scuole, università, tribunali, comparti della pubblica amministrazione in cui le stesse funzioni, le stesse operazioni vengono compiute con costi molto inferiori a quelli di altri; con minori unità di personale, con tempi più rapidi, con servizi migliori. Se è così - e le analisi raccolte nel «Libro verde» sulla spesa pubblica lo confermano senza possibilità di dubbio non c'è ragione per cui non si debba allinearsi verso l'alto, eliminando le inefficienze che gravano sull'intero Paese e che tengono gonfia la spesa. Occorre prendere il modello delle realtà migliori presenti in Italia, premiando l'adeguamento a queste delle meno efficienti. Uno sforzo di riqualificazione della spesa ha interessato tutti i Ministeri. Revisione sistematica del bilancio, riesame delle priorità, analisi dell'efficacia delle politiche e dell'efficienza organizzativa devono diventare parte integrante del servizio che i pubblici uffici rendono al Paese. Non sono mere tecniche di gestione; sono, devono essere, l'atteggiamento mentale di chi sa di amministrare beni non suoi, risorse prodotte con fatica dagli italiani attraverso il loro lavoro. La manovra di bilancio introduce misure di razionalizzazione della spesa per un risparmio complessivo di 4,5 miliardi, pari pari a quasi la metà delle risorse recuperate per sostenere il complesso degli interventi previsti dalla manovra di bilancio. Una parola va detta anche sui cosiddetti costi e spese della politica. Ritengo che gli sprechi quantitativamente maggiori non siano quelli della politica (moralmente i più gravi), bensì quelli del malo uso delle risorse pubbliche nei diversi comparti dell'amministrazione. Per malo uso non intendo la scarsa applicazione al lavoro, i cosiddetti fannulloni, che pure esistono a fianco di tanti impiegati e funzionari coscienziosi. Intendo strutture inutilmente pesanti: troppe Province, troppi uffici, troppi tribunali, lavori svolti magari con scrupolo ma con tecniche superate, o lavori non più necessari. Ciò detto, sprechi e malversazioni nella politica indubbiamente ci sono: sono opera di una minoranza, stranamente tollerata dalla maggioranza dei politici onesti, i quali spesso (si consenta di dirlo a un osservatore che non è un politico di professione), molto più spesso di quanto non si creda, sono impegnati nel compito al quale sono stati chiamati dagli elettori senza risparmio di forze e di passione civile. Sprechi e malversazioni - aggiungo - spesso osservati con pigra indulgenza - al momento del voto - dagli stessi cittadini elettori che se ne lamentano. Una riduzione del personale parapolitico, dei consulenti, delle troppe commissioni di studio è possibile e ormai ineludibile. Il Governo vi si applica da un anno e la persegue anche in questa legge finanziaria, con un complesso di misure che porteranno ad una riduzione della spesa legata alla politica. Nel complesso, si tratta di un'azione vigorosa che porterà un risparmio per le casse delle pubbliche amministrazioni pari a circa un miliardo a regime. Ma c'è di più: nel quadro del disegno di riforma costituzionale che inizierà il suo *iter* tra breve alla Camera, il Governo auspica e sostiene una forte riduzione del numero dei parlamentari sin dalla prossima legislatura,

Sul terreno dell'efficienza - che in un mondo di risorse scarse è requisito primo per poter crescere - il Governo, la politica economica debbono fare ciò che loro compete: nulla di più e nulla di meno. Investire nelle infrastrutture, togliere vincoli e bardature inutili e costose all'attività delle imprese, garantire la sicurezza sul territorio e condizioni fiscali allettanti per gli investitori italiani e stranieri. In relazione con le recenti vicende sui mercati finanziari e con i dati più recenti dell'economia italiana, la manovra di bilancio si fonda su stime di crescita prudenti: poco sotto il 2 per cento quest'anno, 1,5 l'anno prossimo. Per un Governo, sia esso centrale o locale, efficienza significa prima di tutto fornire in modo efficace e al minor costo possibile i beni pubblici primari: legalità, certezza del diritto, sicurezza, correttezza dei comportamenti pubblici. Per stimolare iniziative economiche che producano ricchezza nessuna politica meridionalistica sarebbe più efficace del pieno ritorno di alcune Regioni italiane alla legalità, ad una giustizia certa e rapida, ad un accettabile ordine pubblico. Per ottenerlo occorrono risorse ed il Governo è convinto che esse possano essere innanzitutto tratte da un migliore uso di quelle che già sono in dotazione alle pubbliche amministrazioni. In aggiunta, la manovra di bilancio propone che siano destinate risorse aggiuntive nella misura di oltre 200 milioni per il comparto della sicurezza; per la giustizia, è di particolare rilevo l'iniziativa per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (circa 70 milioni nel prossimo triennio), volto a fronteggiare situazioni di emergenza in questo settore. settore. Scuola: in un mondo di competizione planetaria in cui la produzione di ricchezza è basata sulla conoscenza, l'efficienza si fonda sulla qualità del cosiddetto capitale umano. È urgente che il nostro sistema scolastico colmi il ritardo di cui soffre nel confronto internazionale. Una scuola di qualità inadeguata immiserisce la persona, frena la mobilità sociale e la produttività del Paese. Ecco le considerazioni che hanno indotto i Ministeri dell'istruzione e dell'economia ad un impegno congiunto, che si è tradotto nel "Quaderno bianco sulla scuola", presentato nei giorni scorsi. Tre sono le indicazioni operative del Quaderno: valorizzare la figura dell'insegnante attraverso innovazioni nel reclutamento e nella formazione. Ora, con questa manovra di bilancio si avvia la sperimentazione monitorata di un'azione congiunta tra Stato, Regioni, altri enti locali e istituti scolastici che, a livello di singoli territori, permetta una migliore allocazione delle risorse finanziarie. Dove l'intervento avrà successo, i risparmi realizzati potranno essere reinvestiti a favore dei servizi che si è scelto di potenziare. Università: nelle scorse settimane, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza dei rettori hanno convenuto sulla necessità di elevare la qualità globale del sistema universitario, garantendone la stabilità finanziaria e stabilendo con chiarezza le reciproche responsabilità in un orizzonte temporale che consenta a ciascuna parte di operare con minori incertezze. Mi auguro che sia al più presto firmato un patto per l'università, quale tassello importante di una politica che leghi l'incremento delle risorse fornite dallo Stato attraverso la manovra finanziaria a risultati e miglioramenti nell'organizzazione, nella didattica e nella ricerca, valutati secondo parametri seri e condivisi. Infrastrutture e Mezzogiorno: ammodernare e potenziare le infrastrutture del Paese, recuperare il Mezzogiorno alla economia produttiva sono presupposti fondamentali affinché il nostro sistema economico possa colmare il ritardo di competitività e di crescita rispetto ai principali Paesi europei. Con questa manovra di bilancio il Governo conferma il proprio impegno a dotare il Paese di una rete di infrastrutture al passo con i tempi. Circa due miliardi e mezzo di euro vengono destinati al capitolo investimenti da realizzare nell'anno in corso. Di questi, oltre un miliardo è destinato al gruppo Ferrovie, mentre 215 milioni sono stati stanziati a favore dell'ANAS. Circa un miliardo, infine, è destinato ad interventi per la mobilità a Milano, Roma, Napoli e per il Mose di Venezia; il resto è stato destinato ad investimenti in materiale rotabile nella regione Calabria, al potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina e a interventi di collegamento stradale nella Regione Friuli-Venezia Giulia. A ciò si aggiungono 7 miliardi di euro complessivamente previsti per investimenti in infrastrutture, anche grazie al rifinanziamento delle opere previste dalla legge obiettivo per il triennio 2008-2010, risorse che si aggiungono agli oltre 3 miliardi stanziati nella precedente finanziaria. Ricordo che la media annuale della precedente legislatura è stata di circa 1,8 miliardi di euro. Nel complesso, si perviene ad un importo complessivo destinato alle infrastrutture pari a quasi 35 miliardi di euro. L'effettiva allocazione di tutte queste risorse ai progetti inseriti nei nei principali programmi infrastrutturali è stata accompagnata da una attenta verifica. Il tema Mezzogiorno e sviluppo esemplifica come l'azione di bilancio non trovi il proprio valore soltanto negli indispensabili finanziamenti, ma anche, e talvolta soprattutto, in un più efficace utilizzo delle risorse disponibili. Le nuove risorse connesse all'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, in cui vengono fatti confluire il Fondo per le aree sottoutilizzate e i Fondi europei, sono complessivamente molto significative in particolare per il Mezzogiorno, per cui ammontano ad oltre 100 miliardi euro. Si tratta di una occasione importante, da non sprecare. Di grande rilevanza è anche la riconversione del sistema degli incentivi (legge n. 488) verso meccanismi automatici a sostegno degli investimenti. Fiscalità, semplificazione e riduzione dei costi: alla intensificazione dei controlli deve corrispondere uno sforzo per rendere il sistema fiscale progressivamente più semplice e meno gravoso dal punto di vista degli adempimenti. È importante sottolineare che la semplificazione risponde ad una esigenza fortissima dei contribuenti, in particolare delle imprese. Su questa via la finanziaria compie passi avanti davvero incisivi: propone misure di semplificazione di eccezionale rilievo che non hanno precedenti in molti anni di storia del nostro sistema tributario. La prima innovazione è la predisposizione di un regime speciale per i contribuenti cosiddetti marginali: circa un milione di piccoli imprenditori, con basso giro di affari e senza dipendenti, potrà scegliere di aderire - se lo riterrà conveniente - ad un sistema semplificato con cui assolvere gli obblighi fiscali con un solo prelievo ad aliquota fissa. A sostanziale parità di gettito complessivo per il Fisco, il risparmio in termini di costo degli adempimenti e di tempo impiegato a tenere in regola la documentazione fiscale è enorme. Non meno importanti sono le novità in tema di tassazione per le imprese. Adottando un sistema già sperimentato con successo in Germania, viene semplificata la determinazione della base imponibile facendola sostanzialmente coincidere con il bilancio civilistico: mentre la base imponibile viene allargata, sono abbassate le aliquote di prelievo sia dell'IRES (dal 33 al 27,5 per cento), sia dell'IRAP (dal 4,25 al 3,9 L'IRAP diventa pienamente imposta regionale e viene eliminata dalla dichiarazione dei redditi Unico. Le due misure riducono in modo sostanziale gli oneri per la gestione amministrativa del settore produttivo. Energia e ambiente: così come l'accumulo di un enorme debito, il depauperamento delle risorse naturali è un altra caratteristica con cui si manifesta lo sguardo corto, l'incapacità di allargare il respiro nelle scelte di politica economica. Con la manovra si rafforzano gli interventi per combattere i cambiamenti climatici, per risparmiare energia e migliorare la qualità della vita degli italiani. Tra i maggiori interventi previsti ricordo: la conferma degli stanziamenti del Fondo per Kyoto (600 milioni), la destinazione di oltre 150 milioni alla nascita di nuovi parchi urbani e di ben 530 milioni per combattere il dissesto idrogeologico del Paese; l'estensione degli sgravi fino al 55 per cento per le spese di ristrutturazione delle abitazioni secondo criteri di ecoefficienza (per ridurre le dispersioni termiche e per l'istallazione di pannelli solari) Il risanamento non è certo l'unico fine dell'azione di Governo. Vorrei dire che, a rigore, non è nemmeno un fine in sé; è piuttosto una necessità, un mezzo, una condizione per rendere sostenibile la crescita. Chi rimprovera al Governo e a questa finanziaria di non aver destinato l'intero extragettito al risanamento, non solo si contraddice (perché nelle stesse righe dice anche esattamente l'opposto, che cioè tutto doveva andare alla riduzione delle imposte), ma ignora anche che un Governo non può e non deve omettere il sostegno ai cittadini meno fortunati. Sul terzo indirizzo dell'azione di Governo (terzo solo in ordine di elencazione, non certo in ordine di merito), cioè l'equità, la manovra di bilancio - con i provvedimenti che l'hanno preceduta e con quelli che l'accompagnano nel collegato - contiene una fitta rete di interventi su una pluralità di settori cruciali per la vita della nostra società. Ricordo brevemente alcuni degli interventi che realizzano questa direttrice di fondo. Incapienti: per i soggetti con redditi inferiori al minimo imponibile, un *bonus* di nuova ideazione assicurerà un aiuto concreto, anche se limitato, in tempi brevi. Si tratta di una popolazione di oltre 10 milioni di persone. Il *bonus*, pari a 150 euro per contribuente, è commisurato all'ampiezza dell'eventuale nucleo familiare e sarà perciò corrisposto anche per ciascuno dei familiari a suo carico. Famiglie:si introduce il congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento, effettuando una completa equiparazione a quanto previsto per i figli biologici. Vengono estesi i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo alle vittime del crimine, nonché ai loro familiari superstiti. Donne: prosegue la politica di contrasto della violenza alle donne con un incremento significativo dei fondi destinati a questo scopo. Giovani: si introduce uno sconto fiscale di circa 300 euro l'anno ai giovani tra i venti e i trenta anni che affittano casa e viene ampliato lo sconto per le locazioni degli studenti universitari. Immigrazione: viene incrementato il fondo per l'inclusione sociale. Anche interventi apparentemente di altra natura sono, in realtà, misure di equità. Basti pensare alla condizione dei milioni di pendolari che giornalmente si recano sul luogo del lavoro e troppo spesso soffrono di vero e acuto disagio per capire che l'equità ha anche questa dimensione. Gli investimenti per infrastrutture (ferrovie, strade, metropolitane, altri mezzi pubblici urbani) non potevano attendere oltre e sono stati fortemente incrementati. Questione casa: alla questione della casa il Governo dedica, in questa manovra di bilancio, un insieme organico di misure che non ha precedenti da molte legislature. Dall'ICI agli affitti, dalle abitazioni destinate ai ceti sociali meno favoriti ai giovani che ancora vivono nella famiglia di origine. È urgente la ripresa di una politica per la casa, che incoraggi e premi forme adeguate di edilizia popolare. È quanto il Governo ha iniziato a fare con la costituzione, tramite il demanio, di una società per l'acquisizione, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo. Sono messi a disposizione, per questo scopo, 150 milioni già a partire dall'anno in corso. L'intenzione è di rendere disponibili non meno di 8.000 appartamenti l'anno, per i prossimi dieci anni, a canoni sostenibili, soprattutto nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo. A partire dal 2008 si attua una riduzione permanente del prelievo ICI sulle prime case, a vantaggio dei proprietari che le abitano. Si attuano corrispondenti agevolazioni fiscali a chi abita in affitto. Si tratta, nel complesso, di un intervento di restituzione fiscale molto sostanzioso, pari a circa 2 miliardi di euro a regime. Previdenza: accanto a questa dimensione, volta a ridurre ingiustizie per così dire orizzontali, vi è una seconda dimensione dell'equità, consistente nel contrastare iniquità intergenerazionali, quelle che gravano sulle spalle di chi eredita le scelte del passato. La finanziaria 2008 opera con determinazione in questo campo. Ecco perché la prospettiva di un graduale aumento dell'età pensionabile, in presenza di un allungamento della speranza di vita che è tra gli aspetti più straordinari della nostra epoca, è mantenuta aperta con il recente accordo sulla previdenza, che ha, d'altra parte, giustamente graduato questo aumento superando il brusco e iniquo passaggio, in una sola notte, dai cinquantasette ai sessanta anni per il pensionamento. Ecco perché questa finanziaria e i decreti che l'hanno preceduta e che l'accompagnano hanno scelto di sovvenire alla precarietà dei rapporti di lavoro così da coprire gli intervalli tra un'occupazione e la successiva, in un'epoca nella quale la flessibilità del posto di lavoro è senza alcun dubbio destinata a rimanere molto alta. La manovra comprende le norme che danno attuazione al Protocollo su previdenza, lavoro e competitività firmato lo scorso luglio. Le risorse complessivamente destinate a questo fine sono sostanziose: oltre 5 miliardi di euro per il periodo 2008-2010, che si aggiungono ai 900 milioni di euro per il 2007 e un miliardo e mezzo a decorrere dal 2008 stanziati all'inizio di luglio. In campo previdenziale, il processo di riforma iniziato nei primi anni Novanta viene finalmente portato a un punto che dà certezza ai lavoratori, migliora l'equità - tra e entro le generazioni - delle nostre regole previdenziali e assicura la sostenibilità finanziaria. Lavoro: in tema di lavoro, lo sforzo si è applicato ad accrescere l'efficacia della disciplina del mercato, a incoraggiare una partecipazione semprepiù alta alle forze di lavoro e a offrire tutele adeguate contro il rischio di percorsi lavorativi frammentati. Il Governo propone di riformare il sistema di sostegno alla disoccupazione aumentando la durata e la copertura dell'indennità ordinaria e di quella a requisiti ridotti. Di agire sulla probabilità di inserimento stabile nel mercato del lavoro delle coorti più giovani, delle donne e degli ultracinquantenni attraverso il supporto a iniziative individuali di inserimento che sostengano i redditi dei lavoratori parasubordinati per i periodi d'interruzione. Di potenziare i servizi per l'impiego, collegando e coordinando l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, razionalizzando gli incentivi, aumentando la convenienza di formule contrattuali stabili, contrastando il lavoro nero e tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori. Riteniamo di avere conseguito risultati importanti in questo primo scorcio di legislatura, ma rimaniamo anche convinti che per rendere completo, davvero equo, equilibrato il sistema di protezione sociale italiano, che è ancora insufficiente per molti aspetti, i passi da compiere siano ancora molti; contiamo di compierli. Per quanto riguarda in un mondo che si va unificando, in cui il volto sofferente del nostro prossimo è quello di un africano o di un asiatico che entra nelle nostre case attraverso la televisione, equità e solidarietà sono comandamenti da osservare innanzitutto su scala planetaria. Sempre più attuale appare la previsione formulata nel 1795 da Emanuele Kant: la violazione di un diritto in un punto qualsiasi della terra sarà avvertita come riguardante ciascun uomo. Da noi vi è - per fortuna - soprattutto povertà relativa; la povertà assoluta prevale in altri continenti. L'Italia, Paese ormai prospero nel contesto mondiale, da anni pratica, con beneficio anche per il suo sistema produttivo, la cooperazione allo sviluppo del Sud del mondo. Ma nella passata legislatura, nonostante gli impegni sottoscritti, aveva arrestato la sua azione. Questa è oggi ripresa a sostegno dei Paesi poveri, in particolare nel campo della prevenzione, dei vaccini, della lotta contro le malattie: la manovra che viene oggi presentata destina a questo fine 500 milioni aggiuntivi nel 2007 e 440 milioni nei tre anni successivi. Il Governo è fiero di assolvere questo vero dovere etico e politico e spera di ulteriormente incrementare il contributo nel rispetto di un uso particolarmente attento e oculato delle risorse pubbliche a ciò destinate, quale purtroppo non sempre si è avuto negli anni passati. Signor Presidente, onorevoli senatori, non si devono confondere solidarietà sociale e livello di benessere: troviamo equità anche in comunità umane che languono nella povertà assoluta; osserviamo profonde ingiustizie sociali anche in società opulente. Ma nel nostro mondo industriale e postindustriale di divisione del lavoro e di specializzazione produttiva, gli istituti della solidarietà sociale, che operano essi stessi come strutture organizzate quasi in forma di impresa, si disseccano se non c'è produzione di nuova ricchezza. Sul terreno della politica economica, il Governo di questa legislatura ha perciò posto la ripresa della crescita economica al centro della sua strategia; ha mirato, sì, al risanamento dei conti, ma contemporaneamente anche al recupero di efficienza e di produttività e al sostegno delle categorie più povere della popolazione e delle situazioni più disagiate all'interno del Paese, a cominciare dal Mezzogiorno. Risanamento, sviluppo, equità: tre obiettivi, tre valori che si condizionano reciprocamente. Di questa manovra 2008 si sono già lette valutazioni diverse; una delle più curiose è quella di chi la dichiara una legge elettoralistica. Di solito, questa qualifica vuole dire largo alle spese senza guardare all'equilibrio dei conti, per avere più voti. L'esatto contrario di quanto stiamo facendo: conti in ordine, investimenti per la crescita. Se, però, si vuole dire con questo che la finanziaria risponde alle richieste dei cittadini e, dunque, è suscettibile di creare consensi, allora sì, mi sta bene l'etichetta che fa riferimento all'elettorato. A questa manovra di bilancio hanno cooperato intensamente le diverse anime della coalizione che governa l'Italia, ciascuna portatrice di esigenze reali, fondate, giustificate, vorrei dire, sacrosante, perché tutte radicate in valori, legittimi interessi e attese di cittadini italiani. Fare la sintesi di diverse esigenze costituisce l'essenza stessa del governare; una sintesi che non può mai essere mera sommatoria di richieste, che deve cercare una risposta coerente all'interesse generale, interesse che pur esiste, anche se parla con voce troppo flebile. Questo e non altro è il compito della politica. Se un anno fa mi avessero vaticinato una manovra di bilancio come quella che oggi il Governo propone al Parlamento, non so se l'avrei creduto possibile. Se potremo continuare a svolgere il programma iniziato in questi primi due anni di legislatura, il Paese avrà davvero migliorato il suo volto. Confido che questo sarà riconosciuto, il consenso verrà. Voglio ripeterlo: i fatti sono ostinati e la loro forza alla fine è irresistibile. *(Vivi,

Prima di passare

ieri è avvenuto a Siena un fatto molto grave. Abbiamo tutti letto la notizia della rapina operata da un terrorista, perché non si tratta di *ex* terroristi, ma di terroristi in piena regola, e di fronte a questo episodio, di un detenuto che godeva del regime di semilibertà pur essendo condannato all'ergastolo, un pluriergastolano, abbiamo assistito a dichiarazioni del ministro Amato, il quale affermava che i magistrati devono essere consapevoli di esercitare una responsabilità enorme e credo che lo siano. Ora, di fronte ad un fatto così grave

che sarebbe ancor più necessario che il Governo assumesse, nella sua responsabilità, un provvedimento d'urgenza per sospendere i benefìci della legge Gozzini per taluni tipi di reato.

Presidente, avevo chiesto, a caldo, la parola perché volevo ricordare al collega Calderoli, che tra l'altro è anche Vice presidente del Senato e tutti quanti noi apprezziamo come conoscitore minuzioso del Regolamento,

di un terrorista che non ha mai chiesto scusa a quanti ha creato danno, di un terrorista che era nella direzione strategica delle Brigate Rosse.

del terrorista dice che si trovava in una brutta situazione perché doveva fare il pendolare. Un terrorista era libero e faceva il pendolare. Probabilmente questo terrorista ce l'aveva

in tutti i tavoli dei convegni culturali a spiegare la loro situazione. Davanti ad una situazione del genere, Presidente, credo che i Ministri dell'interno e della giustizia non si possano nascondere dietro un dito solo con dichiarazioni, ma debbano venire in Parlamento a spiegare i motivi per i quali un condannato a tre ergastoli è stato rimesso in libertà e per poco non ha ucciso un agente di polizia che faceva il suo dovere. brevemente perché dobbiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno. STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, il nostro Regolamento ci consente di poter illustrare una questione e credo che mai come in questo caso l'avverbio brevemente sia inappropriato, visto che stiamo parlando - come dicevano i colleghi Gramazio ed Eufemi di una vicenda che ha turbato la pubblica opinione e anziché l'invito alla brevità mi aspetterei dal Presidente del Senato la stigmatizzazione di quanto sta accadendo. Pensare che ciclicamente, vent'anni dopo quella stagione, le pagine dei giornali debbano essere riempite dai nomi dei terroristi che sono in circolazione, credo sia qualcosa di veramente grave.

quella che registriamo in quest'Aula perchè purtroppo non c'è la sensibilità di mandare nessuno dei 103 Ministri, Vice ministri e Sottosegretari quando quest'Aula si riunisce e credo che ciò alquanto scandaloso. Avrebbero potuto immaginare che questa mattina si sarebbe sollevata questa questione, ma l'insensibilità di questo Governo è totale sul fronte delle questioni che più imbarazzano ed indignano i cittadini. Pertanto, le chiedo, Presidente, un'immediata convocazione del Ministro dell'interno per dirci qual è la situazione sul fronte del terrorismo, quanta gentaglia che rischia di assassinare persone e appartenenti alle forze dell'ordine non so se il Ministro dell'interno, nella nota che ha diffuso ieri, fosse colto dal solito candore che lo riguarda ogni volta che avviene un fatto nel nostro Paese. So solo che questa mattina non piangiamo la morte di un altro poliziotto semplicemente perché una pistola era inceppata,

Vogliamo sapere che cosa lo Stato è in condizione di fare per garantire la sicurezza dei cittadini e degli appartenenti alle forze dell'ordine. Presidente, ricordo che mesi fa, insieme al collega Selva, sollevai una questione di indubbia delicatezza: è tollerabile che, in un Paese democratico che dice di contrastare il terrorismo, all'interno del Ministero dell'interno figuri, come porta borse di un Sottosegretario, il terrorista Roberto Del Bello? Siamo stanchi di vedere al Viminale terroristi. Il ministro Amato, prima di parlare di certe questioni, farebbe bene a chiedere al suo Sottosegretario di mettere alla porta un assistente parlamentare condannato all'epoca del delitto Taliercio.

sentire anche il Ministro della giustizia su quella casta privilegiata di magistrati che vanno in aereo e usano le macchine e che molto spesso additano noi come casta privilegiata.

pericolosi, che non fanno il loro dovere e che non meritano spesso di essere loro ancorati a noi nella qualificazione finanziaria, politica ed amministrativa. *(Applausi

sul piano industriale di Alitalia con particolare riguardo all'aeroporto di Malpensa. Ricordo ai colleghi che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Presidente, onorevoli colleghi, per il mandato parlamentare che il popolo padano, che mi onoro di rappresentare, mi ha dato,

fare ludico, bensì costruiva aeroplani. Voglio ricordare che la Provincia di Varese, in particolare, è detta la «Provincia con le ali». Negli anni '20 e '30 correva un detto nel mondo aviatorio italiano per cui «chi mal fa, mal pensa».

tanto che adesso vogliono castigare questo *hub***,** in cui il popolo del Nord ha creduto da sempre operando grandi investimenti. Che il malessere di Roma contro Malpensa è sempre esistito lo vediamo in particolar modo noi fruitori: quando quando arriviamo a Roma da Malpensa veniamo scaricati nel settore B e non nel settore A, come si trattasse di un volo intercontinentale. La cosa, a dir la verità, come padano mi fa anche piacere:

nei comitati organizzativi contro la nascita di Malpensa, che in prima persona si impegnavano a scrivere invitando i comitati a boicottare la nascita del grande aeroporto di Malpensa 2000.

dell'Alitalia; si lavori per confermare la vocazione per cui è nata Malpensa, quella di essere cioè un grande *hub* intercontinentale. Questi sono i due assi, che secondo la nostra opinione possono marciare indipendentemente.

secondo il piano industriale che il presidente dell'Alitalia ha definito di sopravvivenza e transizione. È finalmente una scelta nuova per affrontare la situazione dell'Alitalia. Devo dire che fin qui - lo ricordo, - lo ricordo, perché altrimenti sembra che fino a quindici mesi fa non abbia governato nessuno - gli interventi sono stati assolutamente insufficienti e negativi.

a buttare risorse pubbliche dei cittadini italiani nel calderone, proseguendo una situazione che non era più possibile rimanesse non era più possibile rimanesse in piedi, e infatti non stava e non sta più in piedi. L'innovazione che introduce il Governo è questa; trasformare profondamente nel tentativo di conservare la compagnia

di dati clamorosi che ci dimostrano come, ad esempio, le grandi compagnie europee abbiano una forza straordinaria sul mercato nazionale. Ad esempio, Air France ha oltre il 90 per cento di copertura del mercato nazionale,

ha dato fin qui, perché si esca finalmente dal pantano in cui siamo andati a finire con l'impostazione di questi anni. Nello stesso tempo, pensiamo si possa mantenere

hanno voluto mantenere un ruolo a Linate contro l'alternativa Malpensa, con un aumento dei costi molto forti per l'opera di fideraggio che Alitalia doveva svolgere per portare i passeggeri là:

l'Alitalia verso nuovi azionisti di riferimento che abbiano la capacità e l'intenzione, naturalmente, di rinnovare un impegno finanziario per la compagnia, riproponendone una prospettiva di sviluppo che l'azionista Stato in questo momento non è nelle condizioni di poter garantire. Tale quadro mira al salvataggio della compagnia che arriva in queste condizioni anche per effetto del fallimento della procedura di vendita attivata dal Ministero dell'economia, che il 31 luglio ha dovuto ammettere appunto tale

In questa condizione, il piano di sopravvivenza prevede un restringimento del campo d'azione di Alitalia soltanto nel quadro dell'*hub* intercontinentale di Fiumicino e non dell'altro *hub* intercontinentale di Malpensa. pone dunque una questione Malpensa che va affrontata e risolta.

che quell'*hub* possa e debba servire circa 23 milioni di cittadini italiani, nonché le regioni periferiche di altri Paesi europei che possano confluire e convergere su tale aeroporto. Quindi, il tema delle infrastrutture a terra è centrale e chiediamo un forte impegno del Governo in questa direzione. impegnare il Governo a fare in modo che Alitalia, che possiede oggi circa 350 *slot* che non gli sarebbero più necessari su Malpensa, renda immediatamente disponibili questi *slot* e non utilizzi il e non utilizzi il tempo che Assoclearance le lascerebbe, com'è di rito in questi casi. Vorremmo, anche in virtù dell'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione (che un ruolo alle Regioni in questo senso), vista anche la straordinarietà della quantità di *slot* che si renderebbero disponibili, che le Regioni giochino un ruolo, vengano sentite e possano determinare un'iniziativa nella direzione della riassegnazione degli *slot*. Suggeriamo e impegniamo il Governo a rivisitare con urgenza (questo è un aspetto innovativo per quest'Aula e, in generale, come tema) i trattati bilaterali con gli altri Paesi che avevano come riferimento la tutela della compagnia di bandiera. Non esistendo più la compagnia di bandiera, gli accordi bilaterali con gli altri Paesi possono essere rivisti in funzione degli interessi degli scali aeroportuali.

Da tale mozione, anche per attivare la convergenza della maggioranza,

Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza, perché in un dibattito di questa importanza, che riguarda i trasporti e la mobilità nel nostro Paese,

così importante, delicata e strategica che riguarda non solo migliaia e migliaia di lavoratori del nostro Paese, ma soprattutto il futuro del trasporto aereo, della mobilità, della logistica e di tutto ciò che abbiamo posto all'attenzione del Parlamento. Pertanto, la pregherei, signor Presidente,

perché mi rendo conto che il nostro dibattito deve comunque andare avanti. Abbiamo altri argomenti all'attenzione del Senato altrettanto importanti, però la inviterei, nel rispetto

e che soltanto la politica e la non politica dei trasporti in questi ultimi anni ha portato al semi-fallimento.

non abbiamo ascoltato in questo dibattito qual è la posizione del Governo sul futuro del trasporto nel nostro Paese e in particolare sul trasporto aereo, sulle politiche del cargo, su come intercettare dal Medioriente, dal Mediterraneo non solo passeggeri, ma anche merci, in sinergia con una politica di sussidiarietà tra Malpensa e Fiumicino, per diventare

terminasse senza chiarire che non c'è nessuna concorrenza tra due aeroporti così importanti. La vocazione di Malpensa appare sempre più chiara: una vocazione straordinaria che bisogna potenziare non solo nelle infrastrutture, per rendere sempre più agibile un aeroporto che può diventare un *hub* europeo, in concorrenza magari con altri aeroporti come Francoforte, come Amsterdam, come la stessa Parigi;

se le politiche del Governo sono quelle di mettere sempre, in ogni occasione, sotto pressione, per interessi diversi, Alitalia, che molti amano definire compagnia di bandiera, ma non lo è più, ovviamente Alitalia diventa un punto di di piattaforma sociale in termini di esubero del personale, in termini di non ben precise spese e risorse

quella di dire che la compagnia non è in grado di sostenere due aeroporti, che Alitalia non è in grado di stare a Malpensa e a Fiumicino, che sceglie una strada che è quella di ancorarsi, anche nell'armamento di tutta la flotta, del personale, in un solo *hub* e noi dobbiamo credere che questa ristrutturazione possa essere utile affinché questa compagnia possa diventare privata, che possa diventare punto di riferimento di un solo *hub*, ma soprattutto che Malpensa, che le politiche del Nord, che gli imprenditori del Nord siano aiutati dal Governo a costruire una compagnia del Nord che sia ancorata, dal punto di vista degli interessi, del futuro, del personale, nella parte Nord del Paese. Due grandi compagnie private,

puntuali, a basso costo e possano andare in tutto il mondo. Questo è quello che interessa il Parlamento: le politiche industriali le facciano gli imprenditori, ma soprattutto il Governo alzi la testa e dica quale politica del trasporto, non solo aereo, ma in generale,

Signor Presidente, colleghi senatori, la crisi di Alitalia rappresenta, senza dubbio, una delle vicende più amare della storia delle partecipazioni statali del nostro Paese. È una crisi che deriva dalla somma di una serie di errori politici, gestionali e dai quali nessuno degli schieramenti politici presenti nello scenario nazionale può chiamarsi fuori. Anni di piani industriali sistematicamente disattesi e occasioni perdute di scelte mancate hanno prodotto la situazione drammatica che oggi è sotto gli occhi del Paese e in discussione in quest'Aula. Alitalia ha perso 626 milioni di euro nel 2006, 211 nei primi sei mesi di quest'anno. Ha un indebitamento che, nel 2007, supererà il miliardo di euro. È una compagnia che negli anni Settanta si collocava al settimo posto nel mondo ed oggi è ridotta a dimensioni regionali, con scarse possibilità di sopravvivenza. Poche settimane fa, il consiglio di amministrazione ha varato un piano industriale definito di sopravvivenza e transizione. Ne conosciamo solo le linee guida. È stato criticato sotto molti aspetti, ma parte dalla realtà di una compagnia che oggi mette in campo soltanto 23 velivoli per il lungo raggio su due cosiddetti *hub* che oggi totalizzano 30 milioni di passeggeri a Fiumicino e poco meno di 22 milioni a Malpensa. Il confronto con i competitori europei è impietoso: Air France-KLM possiede 170 aerei a lungo raggio, Lufthansa 134 e British Airways 130. Gli *hub* sui quali ci confrontiamo e su cui gravitano tali grandi compagnie europee, muovono 68 milioni di passeggeri a Londra, 57 milioni a Parigi, 53 milioni a Francoforte, 46 milioni ad Amsterdam,

È finalmente venuto il tempo di lasciare più spazio - il giusto spazio - alle ragioni del mercato, nel momento in cui si discute il futuro di questa compagnia, completando la procedura di vendita, chiudendo la stagione delle interferenze, assumendo tutti (le forze istituzionali, i sindacati) le proprie responsabilità in una fase in cui sono richieste scelte difficili se vogliamo difendere il patrimonio occupazionale industriale rappresentato da Alitalia per il nostro Paese. L'Italia per due motivi non può più permettersi di impegnare ulteriori mezzi finanziari pubblici in questa compagnia. Il primo motivo è la necessità di destinare risorse alle infrastrutture vere, alla scuola, ai centri di ricerca; non possiamo permetterci di ripetere le scelte fatte nel passato per Alitalia. Il secondo è che la presenza di un pagatore di ultima istanza ha sempre impedito di operare scelte dolorose che già in passato erano indispensabili per salvare questa azienda. Alitalia deve, quindi, provare a camminare con le proprie forze e se ce la farà sarà un bene per il nostro Paese. Oggi si discute anche il tema di Malpensa, che è chiaramente legato al destino di Alitalia. Nei giorni scorsi le istituzioni locali lombarde hanno meritoriamente prodotto manifesti per Malpensa ed hanno assunto varie prese di posizione che evidenziano i risultati positivi conseguiti da questo *hub* aeroportuale che è il più puntuale d'Europa, che nel 2007 ha vinto il premio «*Air Cargo of Excellence*» e che, negli anni più recenti, risulta in crescita come volume di traffico e di passeggeri. Dobbiamo, però, ricordare con oggettività quanto sia travagliata la storia di Malpensa. Un aeroporto che nel 2000 muoveva meno di 21 milioni di passeggeri, pari al 22,4 per cento del totale degli aeroporti italiani, che è sceso fino al 17,2 per cento, per poi riprendersi. Tali dati, che è necessario ricordare nel momento in cui si discutono le ragioni e il futuro di Malpensa, esemplificano bene i problemi che questo grande *hub* aeroportuale ha vissuto dalla sua nascita fino ad oggi. Eppure parliamo di un aeroporto che è al centro di un grande bacino di riferimento che produce il 31 per cento del prodotto interno lordo di questo Paese, che raccoglie il 24 per cento delle imprese, fa registrare il 47 per cento delle importazioni e il 41 per cento delle esportazioni nazionali: è il cuore economico e produttivo dell'Italia! Parliamo di un'area in cui si concentrano il 50 per cento dei movimenti, il 47 per cento del traffico passeggeri e il 75 per cento del traffico merci dell'intero Paese. Le istituzioni locali e territoriali devono anch'esse fare la loro parte. È tempo di abbandonare le strumentalizzazioni politiche che abbiamo troppo spesso ascoltato su questa vicenda, perché su Malpensa le responsabilità sono diffuse. Nessuno può chiamarsi fuori. Gli enti territoriali non possono chiamarsi fuori dai ritardi che si sono accumulati nell'accessibilità di quell'aeroporto, dalle scelte effettuate su Linate, dal fatto che altri scali in questi anni sono cresciuti ma spesso hanno fatto concorrenza, in un sistema non coordinato, all'*hub* di Malpensa. La decisione di Alitailia di dimezzare i suoi voli in partenza da Malpensa e la controproposta di Ryanair di fare dello scalo il centro di una rete di voli a basso costo aprono uno scenario complicato sotto il profilo economico e trasportistico. I sostenitori di Alitailia spiegano che la compagnia in fallimento ha il diritto di non cedere gli *slot* che non usa, per poterli poi vendere ad un futuro acquirente della società. Non è chiaro se questa pretesa abbia fondamento giuridico o giustificazioni economiche.

tutte le lamentele di cui è intessuta la cosiddetta questione settentrionale. Malpensa potrebbe diventare la scintilla simbolica da cui si origina un incendio per il quale già si sono radunate molte condizioni. Romano Prodi, che non ha voluto neppure ricevere il governatore Roberto Formigoni per discutere le scelte della compagnia, che ora è sotto il controllo del suo Governo come quindici anni fa era di proprietà della sua IRI, non sembra rendersi conto della gravità della situazione che si può creare. L'immagine di una grande infrastruttura del Nord, dove di infrastrutture c'è grave carenza, ridotta alla paralisi dalle omissioni o dalle decisioni punitive «romane», può diventare rovinosa. Se è vero, come ha detto il ministro Bersani, che un'azienda sull'orlo del fallimento non può assicurare il futuro di Malpensa, bisogna che non insista nel trascinarla con sé nel baratro. Una nuova e diversa prospettiva per Malpensa dipende naturalmente anche delle scelte di Alitalia. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la sorte del piano di sopravvivenza e di transizione e, soprattutto, del procedimento di privatizzazione della compagnia I temi su cui confrontarsi sono i seguenti: una posizione netta sulla crisi di Alitalia, che guardi agli interessi del Paese; il tema della riorganizzazione del traffico aereo; infine, una piena assunzione di responsabilità da parte del Governo in questa delicata vicenda. «Alitalia non è in grado strutturalmente ed economicamente di supportare l'alimentazione di due *hub*»: è quanto ha sottolineato il presidente di Alitalia, Maurizio Prato, illustrando alla Commissione lavori pubblici del Senato i motivi per cui la compagnia ha deciso di trasferire i collegamenti di lungo raggio da Malpensa a Fiumicino. In particolare, l'attività di feederaggio sull'*hub* lombardo "comporta una duplicazione di costi" che pesano per 150-200 milioni di euro; «i voli di feederaggio viaggiano semivuoti e ripartono vuoti da Malpensa». È evidente - ha argomentato Prato - che «un'azienda sana non lascerebbe un aeroporto come Malpensa, ma non è questo il caso di Alitalia» che è «all'anticamera di una situazione fallimentare», versa in uno «stato comatoso, si trova in camera di rianimazione» e che «non si può permettere di mantenere delle linee in perdita». Quanto a un in perdita». Quanto a un nuovo intervento finanziario dello Stato per salvare Alitalia, si tratta di una strada assolutamente "impercorribile". Per Prato «il difetto» dei diversi tentativi di salvataggio dell'aviolinea è stato proprio quello di essere stati «interventi di natura solo finanziaria». A questo si aggiunge poi il fatto di aver creduto di risolvere i problemi di Alitalia «chiedendo la testa dell'amministratore delegato per ricominciare da capo ogni volta». Entro la prima decade di ottobre Prato conta invece di riferire al consiglio di amministrazione sull'esito del primo *scouting* sui possibili acquirenti della compagnia. Va detto che nel frattempo Ryanair, nella sua offerta, ricalca la decisione di Alitalia di sviluppare i voli a medio raggio, e non gli intercontinentali, e non vede Linate come concorrenziale, mentre Malpensa, dal 2000, ha perso tre punti percentuali di traffico, e Bergamo-Orio al Serio ha quasi recuperato questa perdita. L'idea di fare dell'aeroporto di Varese un *hub* non pare realistica, stante i problemi di collegamento. Uno studio proposto da Ambrosetti mette in evidenza come Malpensa, dopo anni di mal gestione, vede i principali suoi fruitori, gli industriali del Nord, dichiarare di non utilizzare da tempo né Malpensa né Alitalia, «in quanto i collegamenti con i due aeroporti comportano tempi di percorrenza di tre ore in autostrada un'ora c'è l'aeroporto di Verona o Bergamo o Brescia che ti collega a Francoforte e da lì si parte per la Cina o l'India comodamente», volando Lufthansa, ovviamente. Il paradosso Malpensa, inteso come fenomenologia degli errori all'italiana, è anche questo: il *boom* dell'aeroporto sotto casa. Basta l'elenco: Malpensa, Linate, Orio al Serio, Brescia Montichiari, Verona, con distanze di nemmeno cento chilometri l'uno dall'altro; senza dimenticare il resto: Venezia, Treviso, Trieste a Est, Torino ad Ovest; e ancora: Genova, Bologna, Forlì, Rimini. Sarà anche un bacino da 110 milioni di passeggeri, come documenta Ambrosetti, ma è difficile negare che le battaglie, spesso di campanile, per accaparrarsi *low cost* od offrire scali di feederaggio a grandi compagnie inevitabilmente hanno contribuito a cannibalizzare Malpensa che, di suo, con i suoi scarsi e poco veloci collegamenti via treno e auto, ha fatto di tutto per dare spazio alla concorrenza di Lufthansa o Air France per le quali l'Italia è ormai il secondo mercato, senza tener conto che più del 60 per cento dei passeggeri di Malpensa, come ha dichiarato il ministro Bersani, provengono dal Centro-Sud d'Italia.

meglio che Alitalia abbandoni Malpensa, che si dia spazio ad altri operatori e magari si migliorino i servizi di terra. Da tutta questa vicenda, però, gli assenti sono i grandi imprenditori del Nord, che lamentano in continuazione la carenza di infrastrutture; ma nessuno che si faccia avanti, perché il *business* del trasporto aereo forse troppo rischioso anche per loro. Signor Presidente, penso che Malpensa diventi, in qualche modo, emblematica della cosiddetta questione del Nord in quanto una grande potenzialità di sviluppo economico rimane penalizzata dalle difficoltà degli investimenti infrastrutturali e dalle lentezze della politica, delle istituzioni, delle risposte adeguate che devono venire. devono venire. Non sono fra coloro che si ascrivono al partito del Nord e penso che anche la "questione del Nord" non debba essere ristretta ad un'autoreferenzialità o ad uno *slogan* elettorale.

alla consapevolezza delle nostre responsabilità. Penso a tutti i livelli della politica del Paese, ai livelli istituzionali, della Regione e al livello locale. Vi sono questioni, onorevoli colleghi, che non è che necessariamente debbano essere di centro-destra o di centro-sinistra

Su Malpensa e su Alitalia lavorano da anni Parlamenti, amministrazioni di centro-destra e centro-sinistra con colpe, con qualche merito, ma soprattutto con qualche responsabilità. Ebbene, in tutti questi anni in cui i destini di Malpensa e di Alitalia si sono così profondamente intrecciati, oggi è arrivato il momento del *redde rationem*, il momento in cui questi destini intrecciati hanno creato difficoltà ad Alitalia e di conseguenza anche a Malpensa.

(chi frequenta le tangenziali milanesi sa come talvolta sia complesso raggiungere l'aeroporto di Malpensa e sa che quindi in quel settore occorre investire tanto),

Si è al centro dei corridoi più importanti del traffico sia merci che passeggeri. Quindi, è innegabile pensare che Malpensa sia in qualche modo al centro del traffico aereo europeo e non si può prescindere da tale valutazione.

Rivalutando in questa logica il piano industriale di Alitalia, è difficile immaginare e comprendere come mai Alitalia abbia concentrato e stia concentrando tutti gli sforzi di rilancio e di valorizzazione dei propri *asset* su Fiumicino, quando invece la gran parte del traffico e dell'appetibilità anche commerciale si concentra su Malpensa. Se avessi una compagnia aerea piccola e dovessi venderla probabilmente concentrerei i miei sforzi di piano industriale

tutti gli sforzi su Fiumicino, probabilmente dovrebbe anche lasciare liberi il più velocemente possibile gli *slot* di Malpensa, perché se il "risanamento" o la vendita di Alitalia dovesse tardare, e non si libera lo spazio su Malpensa, inevitabilmente la crisi di Alitalia rischia - anzi già sta accadendo - di trascinare anche Malpensa in una crisi di incertezza politica e strategica, che potrebbe creare pesantissime ricadute

o Alitalia rivede il suo piano industriale e valorizza Malpensa, e però si procede velocemente alla vendita della partecipazione statale, in modo che Malpensa possa ritrovare una sua strategia in questa operazione di piano industriale e di vendita, oppure Alitalia faccia un piano più modesto - come sta facendo - di ripiegamento, meno ambizioso, ma lasci libera in qualche modo Malpensa, perché oggi c'è una situazione pasticciata che non va né in un senso né nell'altro, e crea solo incertezza. Penso quindi che il Governo, oltre a procedere nella direzione che sto dicendo, debba anche individuare un tavolo preciso con la Regione Lombardia sul destino degli aeroporti lombardi e che Malpensa trovi la sua ragione anche di pieno sviluppo dentro la riorganizzazione del sistema aeroportuale lombardo, dove ciascun aeroporto scelga la sua vocazione, per evitare sovrapposizioni e conflittualità,

Penso invece che tutti gli aeroporti del Nord possano contribuire, in un sistema anche di programmazione nazionale, a fare sinergie e a garantire il meglio, ad aumentare la ricchezza in quella Regione d'Italia. Favorire gli scambi e lo sviluppo economico penso che significhi arricchire tutta l'Italia, e infine anche dare maggior senso alla funzione di Fiumicino. Quindi ritengo che ci debba essere una grande collaborazione in questo momento di tutti i livelli istituzionali, del Governo e della Regione Lombardia, per trovare una soluzione. Dobbiamo dire che Malpensa deve rimanere *hub*? Certo, questo mi pare sia nelle cose: non è sufficiente dirlo. Le enunciazioni non sono sufficienti né all'aeroporto di Malpensa, né ai cittadini lombardi, né a quelli del Nord, né in generale a tutti quelli italiani; penso che attorno a Malpensa la politica debba dimostrare di saper prendere decisioni veloci, utili allo sviluppo. Pertanto, non è sufficiente fermarci alle enunciazioni, ma bisogna cominciare a lavorare in modo assolutamente concertato fra i diversi livelli istituzionali per il bene del nostro Paese.

colleghi, rappresentante del Governo, grave è la situazione di Alitalia e altrettanto grave è la situazione di Malpensa. La prima, sull'orlo del fallimento, presenta un piano industriale definito di sopravvivenza/transizione, che cerca le condizioni per la prosecuzione dell'attività, ma mette a rischio molti, molti posti di lavoro. La seconda vede ridimensionato il numero dei voli e induce, rende forte la preoccupazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che temono ripercussioni occupazionali entro il sedime aeroportuale e sull'indotto economico, molto rilevante, che ci vive attorno. Questa situazione ha responsabilità ben precise; scelte sbagliate e miopi, incapacità di gestione, inefficienze e sprechi sono tutti riconducibili ai Governi di centro-destra, regionale, provinciale, comunale e, ovviamente, nazionale. Scelte e comportamenti tutti interni alla logica di realizzare a Malpensa un aeroporto *hub* a tutti i costi, ci stia o non ci stia, con o senza Fiumicino. E perché ciò avvenisse, occorreva che Alitalia scegliesse Malpensa a scapito di Fiumicino o alimentasse due *hub* contemporaneamente. Se poi non ce l'avesse fatta o fosse andata in rosso, anche a prescindere dalla cattiva gestione, pazienza, ci avrebbe pensato il Ministero del Tesoro. L'importante era che Malpensa crescesse, si facesse la terza pista, si muovessero gli affari. Oggi è un momento difficile, una fase complessa; ma difficoltà e complessità non possono non costituire, devono costituire un'occasione utile per una svolta, per correggere gli errori del passato e impostare uno sviluppo equilibrato, programmato e coordinato a livello nazionale. Nel progetto Malpensa 2000 è stata investita un'ingente quantità di risorse pubbliche, ma secondo un'impostazione che non teneva conto della realtà di un sistema aeroportuale diffuso, come quello presente nel nostro Paese, che conta oltre 100 aeroporti e in cui l'*hub* di Malpensa ha avuto già da subito difficoltà a esercitare la propria funzione. Non solo; la situazione è stata aggravata al Nord da una mancata e insoddisfacente definizione dei ruoli dei due aeroporti che insistono sull'area milanese e da una politica regionale degli insediamenti disorganica. Il risultato è che oggi, nella vasta area territoriale che dovrebbe insistere su Malpensa, sono insediati aeroporti in rapporto di uno ogni 50 La politica su Malpensa è stata caratterizzata anche dalla deregolamentazione del mercato del lavoro e dalla precarizzazione, dall'incuria e dall'indifferenza per il territorio e l'ambiente, dalla commistione tra affari e politica, da pesanti ritardi nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'accesso e il collegamento con l'aeroporto. Per affrontare in positivo la crisi di Alitalia e Malpensa occorre fuoriuscire dall'impostazione adottata nel passato e respingere nettamente la contrapposizione di tipo ideologico e campanilistico che si tenta ancora oggi - forse forse più di ieri, e in modo ancora più nervoso e aggressivo - di alimentare; contrapposizione di Malpensa nei confronti di Fiumicino, di Milano contro Roma, del Nord contro il Sud, della destra contro la sinistra. In questa fase diventa indispensabile l'accelerazione dei lavori qui in Parlamento sulla legge delega di riforma del trasporto aereo che deve classificare e orientare le funzioni degli aeroporti italiani, la definizione del Piano degli aeroporti in un'ottica di sviluppo razionale di tutto il sistema aeroportuale, entro il quale affrontare la questione degli aeroporti del Nord e prevedere un ruolo definito per Malpensa, che ne sviluppi le potenzialità, indipendentemente dalle strategie di Alitalia e compatibilmente con la sostenibilità del territorio, completando nello stesso tempo gli interventi infrastrutturali necessari. Siamo di fronte a un'occasione importante per impostare uno sviluppo equilibrato e correggere gli errori del passato, ripeto, di cui non devono essere il territorio e i lavoratori a pagare le conseguenze. Malpensa è nata su un tacito scambio, in base al quale i cittadini e le istituzioni locali ci avrebbero rimesso qualcosa a livello di ambiente e di salvaguardia del territorio, ma ci avrebbero guadagnato in occupazione e rilancio dell'economia. Allo stato attuale, però, i costi prevalgono sui benefici: costi ambientali, come l'inquinamento acustico e l'inquinamento dell'aria, lo sbancamento di aree verdi in un territorio prestigioso e indispensabile come quello del parco del Ticino; costi logistici, come il traffico insostenibile del nord della Provincia di Milano, del sud della Provincia di Varese e del Piemonte confinante; costi economici pesanti. Per correggere e non aggravare questi aspetti resta ferma la necessità del ricorso alla Valutazione ambientale strategica, non solo come atto dovuto alla direttiva europea, ma perché sia determinato in modo scientifico il grado di sopportabilità del territorio. Ritengo sia stato un grave errore il diniego della Regione Lombardia opposto ai Comuni e al Parco del Ticino di effettuazione della VAS, che avrebbe consentito di rassicurare le popolazioni e potuto imprimere uno sviluppo più solido ed equilibrato all'insediamento aeroportuale. Ognuno dunque deve fare la sua parte, senza confusione o sovrapposizioni di ruoli ed interessi: il Governo faccia il Governo, la Regione faccia la Regione, il Comune di Milano faccia il Comune. La Regione Lombardia, invece di proporsi come Stato sovrano, si assuma le proprie responsabilità per essersi mossa senza una strategia sul sistema aeroportuale del Nord, per aver tollerato eccessivi ritardi nella realizzazione delle infrastrutture, per non aver salvaguardato l'ambiente, trovato soluzioni idonee per l'indotto, assicurato la qualità dei posti di lavori. La mozione proposta dall'Unione ha il merito di fornire precise indicazioni al Governo, di considerare Malpensa un problema e insieme una risorsa nazionale e di chiamare le istituzioni della Regione Lombardia e dell'area di Malpensa, le forze economiche e sociali a portare un loro peculiare contributo per definire il ruolo di Malpensa in una prospettiva di sviluppo equilibrato, ordinato e moderno.

e primo fra tutti al Presidente della Giunta regionale lombarda, Formigoni, che un aeroporto, anche un grande aeroporto di rilevante interesse locale e nazionale, è pur tuttavia, nella sostanza, un impianto industriale che produce trasporto aereo. Come in un qualsiasi impianto industriale, se nessuno vi porta la materia prima e nessuna porta via il prodotto, l'impianto non produce reddito. Per questo bisogna guardare alla questione di Malpensa come ad una crisi industriale, che è innanzitutto una crisi di impresa; poi ci sono anche le provvidenze pubbliche, non si può scambiare la causa con l'effetto. Le provvidenze pubbliche servono per aiutare una politica di ripresa, ma la politica di ripresa deve derivare dalle scelte dei *manager* della direzione, di quelli che in sostanza hanno la proprietà, le mani in pasta, dell'impianto aeroportuale. Per sapere come possiamo muoverci, bisogna rispondere a due domande. La crisi dell'Alitalia acuisce questa crisi specifica di Malpensa come attività di industria? Sì; la acuisce perché naturalmente viene a mancare un soggetto che opera proprio sul terreno dell'immissione di materia prima e del trasferimento di prodotti lavorati. La ripresa di Alitalia, il suo salvataggio contribuisce alla soluzione strutturale dei problemi di Malpensa? La risposta è no. I problemi di Malpensa sono così profondi che non possono essere risolti dalla sola compagnia di bandiera. La via deve essere un'altra, e cercherò di suggerirla. Nel frattempo però alcuni luoghi comuni debbono essere sfatati per capire come ci possiamo muovere. Per quanto riguarda il primo, il mercato del trasporto aereo italiano è il più aperto alla concorrenza nell'insieme dei Paesi europei. In Francia, Air France ha il 94 per cento del mercato domestico e ha intrapreso e vinto azioni giudiziarie verso aeroporti serviti da vettori *low cost* attraverso contributi all'accesso. In Germania, Lufthansa ha il 68 per cento del mercato domestico e ha acquisito, come propri, vettori *low cost*, acquisito l'intera Swissair, il 10 per cento della società di gestione dell'aeroporto di Francoforte e un *terminal* molto importante a Monaco. Tutte cose che in Italia non esistono.

e gestisce il nuovo *terminal* di Madrid. Alitalia detiene solo il 42 per cento del mercato domestico e non ha ancora concluso l'aggiudicazione di Volare, la quale avrebbe solo il 2 per cento del traffico. Voglio dire ai colleghi della Lega di rammentare che il presidente di Malpensa è quel Bonomi

AZ Alitalia ha il fucile spianato dell'Antitrust. Siamo passati da una fase di monopolio di stato alla liberalizzazione selvaggia e, come spesso accade in questi casi, i *parvenus* del liberismo ultimi arrivati al nuovo credo sono ansiosissimi di dimostrarsi i più zelanti. Questa è una delle cause principali della crisi di Alitalia e di Malpensa. I principali competitori europei sono penetrati ampiamente nel mercato italiano e hanno generato un effetto aspirapolvere da Malpensa verso gli altri *hub* europei. Pensate che Lufthansa e Air France, separatamente, offrono più posti dal mercato italiano ai loro *hub* di Francoforte, Monaco e Parigi. Ciascuno di questi *hub* è servito dalle compagnie straniere che partono dal mercato italiano in misura maggiore di quanto offra, con copertura di posti più limitata, Alitalia da Malpensa.

11,1 milioni di passeggeri all'anno dal Nord Italia, 13,3 milioni di passeggeri all'anno dal Centro-Sud. Questa è la realtà del mercato italiano. Anche il mercato intercontinentale, che costa, vede Milano in posizione arretrata: 2,6 milioni di passeggeri all'anno contro 3,3 milioni di passeggeri all'anno da Roma;

È vero che il traffico *business* ha un'incidenza da Milano del 14,6 per cento migliore di quella di Roma, ma questa incidenza è di quattro punti inferiore alla media di tutti i Paesi europei, fatta eccezione per la Spagna. Alitalia non vola sul lungo raggio intercontinentale, e questo rende molto meno competitivo il federaggio dei voli domestici internazionali. Portare passeggeri a Malpensa è per Alitalia una perdita secca. Opera con 23 aerei contro i 148 di Air France; opera 142 voli settimanali da *hub* contro i 954 di Air France; raggiunge 17 destinazioni dall'*hub* contro le 101 di Air France. Alitalia non riesce ad alimentare compiutamente un solo *hub* e opera, invece, su tre aeroporti principali: Fiumicino, Malpensa e Linate. Due di questi aeroporti insistono sullo stesso bacino di traffico e costringono Alitalia a duplicare i voli sui due aeroporti milanesi, solo per alimentare la rete. Il modello di *network*, come si dice, il modello di rete è antieconomico ed illogico: da Linate partono ben sette rotte internazionali, sottraendole a Malpensa, che è collegata da Alitalia con 54 rotte internazionali e 17 rotte intercontinentali. non è che non ci sono voli da Malpensa: non ci sono i passeggeri*.* Sei passeggeri su dieci

alimentano gli *hub* di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Madrid. Malpensa non è attrattiva per il Nord, nonostante i voli diretti di Alitalia. Di questa situazione, Presidente, occorrerà tenere conto nell'indicare le soluzioni per questo aeroporto.

Vivo all'ombra della torre di controllo di Malpensa, dunque conosco bene la situazione, sono un pilota sportivo

Ecco allora la soddisfazione di andare a Londra per 30 euro e poi, da lì, andare a New York o in giro per il mondo con le compagnie di bandiera di altri Paesi, perché il nostro Governo non ha un'attenzione precisa nei confronti delle compagnie *low cost* nostre concorrenti.

il presidente delle Camere di commercio Sangalli e Bonomi si piangono addosso, mi viene da dire alla Bossi che questi non ce l'hanno duro. Forse è venuto il momento che la Padania si faccia la sua compagnia di bandiera.

gli industriali, il Governatore e il Sindaco di Milano. Mi capita spesso di trovare all'aeroporto di Fiumicino e di Malpensa aeromobili con la scritta «Air Berlino»; non riesco a capire perché, se la città di Berlino ha la sua compagnia di bandiera, non può avere la sua compagnia di bandiera il Comune di Milano, che sicuramente

facilissima: tutti i dipendenti dell'Alitalia godono di voli intercontinentali a bassissimo prezzo, pagando solo il prezzo dell'assicurazione dell'aeromobile, e si fanno le vacanze in giro per il mondo a spese del Nord, che continua a lavorare e continua a pagare, e quando chiede di avere un *hub* per portare avanti i suoi *business* economici per il Paese viene ancora una volta mortificato.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, al centro del dibattito odierno non c'è una battaglia a difesa di interessi campanilistici, non c'è la rievocazione non c'è la rievocazione di un dualismo Malpensa-Fiumicino, che appassiona sempre meno, ma c'è più articolatamente il domani del sistema Italia. Suscitano molteplici perplessità le linee guida del Piano industriale 2008-2010 approvate dal consiglio di amministrazione di Alitalia in data 30 agosto 2007. Discutibili sono i contenuti, che fin dalle premesse, vengono emblematicamente definiti "misure atte a garantire la sopravvivenza e la transizione" di un'azienda, diventata ormai nell'immaginario collettivo come la nazionale di calcio, dove 58 milioni di tifosi sono da un lato pronti a sostituire l'allenatore per risolvere la crisi di risultati, che evidenziano una perdita e non da oggi di un milione e mezzo di euro al giorno, e dall'altro a ritenere che tra le soluzioni più gettonate possa esserci il... "lasciamola fallire". La strategia ipotizzata, dunque, e riferita ad un ridimensionamento della rete di collegamento che gravita attorno a Malpensa, non solo non serve a rilanciare la compagnia nell'Olimpo delle linee aeree, perché intende unicamente salvare il salvabile, ma tende a produrre, laddove venisse attuata, profonde modifiche nella strategia aziendale e dannose ripercussioni sul sistema di trasporto aereo nazionale. Ogni serio ragionamento non può prescindere da alcuni dati di fatto, che ripercorrerò con ordine: l'Alitalia ha una flotta molto dimensionata rispetto ai suoi concorrenti: dati AEA del 2005 rilevano che dispone di 182 aerei senza acquisti all'orizzonte, mentre la Lufthansa ne ha 409 (e 34 già ordinati), l'Air France 253 (37 in arrivo), la British Airways, 289 (10 già prenotati). Dunque, vale ricordare che sotto la sigla AZ si nasconde un topolino che ha approfittato degli aiuti di Stato (5 miliardi di euro in dieci anni) e che l'Unione Europea ha permesso solo a patto che non fossero destinati al finanziamento di nuovi investimenti. Continuando l'analisi dei dati e delle comparazioni utili a verificare la strategia aziendale di Alitalia, che intende nella fattispecie tagliare 150 voli internazionali da Malpensa, non si può prescindere dall'area allargata entro la quale è ubicato tale aeroporto. Essa comprende i territori di Varese, Milano, Como, Novara e Verbania, un'area nella quale è presente una delle più importanti agglomerazioni italiane di persone e di imprese. In un raggio inferiore a 100 chilometri si concentrano oltre 5,5 milioni di persone, a cui si dovrebbero aggiungere i circa 300.000 del Canton Ticino, con una presenza di 75.000 imprese manifatturiere e 697.000 occupati. Con il bacino più esteso (Lombardia, Piemonte, Liguria) si raggiungono 15 milioni di abitanti, 187.000 imprese manifatturiere e 1 milione e 865.000 occupati. È questo uno dei più interessanti bacini europei di consumo ad elevato reddito e di concentrazione imprenditoriale, da cui partono circa 132 miliardi di euro di esportazioni verso il resto del mondo.

Vale la pena ricordare che da gennaio a luglio 2007 Malpensa ha registrato un incremento di passeggeri del 9,2 per cento, *trend* di crescita che consentirebbe di passare

Il valore delle merci esportate dalle imprese lombarde nel corso del 2006 ha registrato un aumento del 9 per cento, passando da 85.277 milioni a 92.910 milioni di euro, valore pari al 28,4 per cento del totale delle esportazioni italiane. Qualora, dunque, le linee di intervento prospettate da Alitalia venissero attuate, risulterebbe evidente la volontà sia di rinunciare a competere con i grandi vettori europei ed internazionali che di allontanare l'Italia, e in modo particolare il Nord, dai traffici economici mondiali. Da questi dati affiora allora ben più di qualche ragionevole dubbio circa la credibilità delle indicazioni contenute nel piano Alitalia, il quale, anziché puntare al rilancio della Compagnia attraverso azioni in grado di recuperare competitività industriale, finirà per comprimerne le potenzialità proprio in ragione del preannunciato abbandono delle rotte intercontinentali che fanno capo a Malpensa. Tali decisioni non sembrano tenere in alcun conto le esigenze di mobilità di quanti operano nelle imprese del Settentrione, che si vedranno allungare i tempi di percorrenza per raggiungere le destinazioni intercontinentali. È stata stimata una dilatazione fino a due ore e mezzo

Non capiamo pertanto come mai persino tra le pieghe del DPEF 2007-2011 esistono risorse destinate a potenziare le infrastrutture intorno a Malpensa e poi si procede in questa direzione. Riteniamo che il Ministero dell'economia, che detiene il 49 per cento delle azioni Alitalia non può limitarsi a spingere per l'eutanasia dell'aviolinea. Se non vuole pronunciarsi sul piano industriale di Alitalia, dica almeno una parola chiara e definitiva per fare in modo che vi sia il coinvolgimento delle Regioni nell'assegnazione degli *slot*, delle rotte e delle bande orarie.

Faccia fronte il Governo alle sue responsabilità, che non sono soltanto quelle di detenere una importante quota azionaria di Alitalia, ma difendere l'intero sistema Italia. Chiarisca che non si tratta di un braccio di ferro tra Nord e Sud! esca da questo assordante silenzio che danneggia pesantemente l'economia dell'intero Paese. Sono sicuro che l'aeroporto di Malpensa, attraverso le azioni del Nord, saprà essere rilanciato in modo da essere competitivo e sicuramente se ne vedranno le conseguenze.

rispetto al calendario previsto, rischiamo di non concludere l'esame della mozione con la conseguente votazione. Ricordo a tutti che la seduta si concluderà alle ore 13,30.

serio e non costituisse un problema strategico di politica economica e di politica settoriale, dei trasporti, trasporti, della logistica, di strategia di crescita di un Paese, potremmo cavarcela con qualche battuta, come ho sentito fare nel dibattito di questa mattina. Potremmo far nascere o incentivare una «Air Padania» o una «Moratti Airlines» e avremmo risolto il problema.

si è sempre e pensato di fare gli interventi e le politiche senza un'idea di piano e senza una strategia. Da questo punto di vista, Malpensa, ma non solo (Malpensa è un fatto rilevante e importantissimo), è il frutto di una politica dei trasporti senza programmazione.

Non basta questo per localizzare un aeroporto a prescindere, come avrebbe detto Totò, dalle politiche dei trasporti, dalle politiche del settore aeronautico, dai rapporti, nella politica dei trasporti, dell'Italia con gli altri Paesi europei. europei. Ci si è imbarcati in un'operazione che non ha né capo, né coda: solo questa modalità d'intervento sulle opere pubbliche sganciate dai piani di settore

sono si mettono in queste condizioni. L'Alitalia è stata messa nella condizione di operare strutturata su due *hub*, un assurdo; non c'è una compagnia

È un assurdo che si spiega con il politicismo, il localismo, il campanilismo, l'approssimazione con cui sono state fatte quelle scelte, per cui oggi Malpensa e Alitalia, nei loro rapporti, si fanno reciprocamente male. Da questo punto di vista, è assurda e stravagante la posizione di tanti liberisti, che ho sentito riecheggiare anche oggi, che a fronte della crisi di Malpensa pensano che che essa si salvi, che si possa rilanciare attraverso la cannibalizzazione di Alitalia; non si salva nessuno in questi termini: dobbiamo essere consapevoli di questo.

come siamo arrivati a questo punto, perché lo scarico di responsabilità può essere divertente dal punto di vista politico, ma non ci porta da nessuna parte; bisogna cominciare a chiedere chi ha fatto quelle scelte e chi le ha fatte dovrebbe risponderne,

diversa natura. Il centro-destra ha le sue dirette e pesanti responsabilità; non lo dico per scaricare quelle che oggi sono a carico di questo Governo, ma per dire che se vogliamo affrontare i problemi

in termini di *cargo*, in termini di voli *low cost*, in termini, forse, di raccordo, di intese internazionali tra Alitalia e altre compagnie anche per le rotte intercontinentali;

Tra l'altro, Alitalia è stata sovraccaricata dei costi di due *hub*. Il personale di Alitalia - lo voglio dire al collega

In questo processo di cosiddetto salvataggio dell'Alitalia, i lavoratori hanno pagato e continuano a pagare in termini di occupazione e di condizioni di lavoro. L'Alitalia Team è la prova più evidente di tutto questo. Se confrontiamo le condizioni del personale operativo di Alitalia con quelle delle altre compagnie, vediamo che il confronto regge alla grande. Dove non regge? Dove non regge? Se confrontiamo le strutture di direzione e di amministrazione di Alitalia, che con tutti i Governi di centro‑destra e di centro-sinistra hanno mantenuto le loro condizioni

Lo chiedo al Governo. Sarebbe cosa utile, proprio nella ricerca di una soluzione per attuare il piano Alitalia, intanto sospendere il titolo dalla Borsa ed evitare, come è successo in passato, che i soldi della ricapitalizzazione venissero bruciati in nome della ideologia della privatizzazione e finissero, in buona sostanza, anche nelle tasche dei gruppi dirigenti di Alitalia,

Roma-Milano, ma riteniamo che un confronto adulto sul delicato tema Alitalia-Malpensa non possa prescindere dalla grande importanza che riveste l'*hub* milanese non solo per l'economia lombarda e non solo per quella del Nord-Italia, ma per l'intero Paese. Noi pensiamo che la materia vada affrontata considerando sicuramente la penosa situazione della compagnia di bandiera, di Alitalia, ma anche il destino dei due principali aeroporti di Fiumicino e di Malpensa, oltre che il sistema complessivo del trasporto aereo italiano e la connessione con le altre modalità di trasporto. Alitalia ha perso 625 milioni di euro nel 2006, vale a dire 1,7 milioni di euro al giorno; il 2007 non sembra molto diverso. L'organizzazione, però (meglio sarebbe dire «la disorganizzazione»), di Alitalia produce disfunzioni gestionali tali da rendere in molti casi antieconomico anche volare a pieno parco: sembra impossibile, però è francamente così. Diversi lustri di decisioni mai assunte, una politica di alleanza a tratti vergognosa, l'uso improprio di denaro pubblico per ripianare debiti pregressi: tutto ciò ha condotto Alitalia sulla strada del non ritorno. È evidente come in queste condizioni (sottolineo: in queste condizioni) Alitalia non possa alimentare due aeroporti come Fiumicino e Malpensa. A questo punto, la cura può essere una sola: vendere Alitalia consentendole di inserirsi in un quadro di alleanze forti a livello internazionale. Auspichiamo l'acquisizione da parte di un grande vettore che operi già attraverso un modello multi-*hub* e che inserisca il vettore Alitalia in una delle tre grandi alleanze mondiali. Il piano industriale di Alitalia concentra su Fiumicino il traffico intercontinentale, ovviamente a nocumento di Malpensa. Eppure, se si fosse intervenuti qualche anno fa, tamponando la crisi di Alitalia e rafforzando la sua politica industriale sia su Roma, sia su Malpensa, differenziando ovviamente anche le tipicità dei due aeroporti, oggi non saremmo in queste condizioni; oggi non assisteremmo alla rinuncia di 150 voli da e per Malpensa, e gli *slot* hanno - come ben sappiamo e come è stato ricordato - un notevole valore economico e commerciale. Allora, vista la decisione inserita nel piano industriale di Alitalia, è indispensabile che questi *slot* vengano immediatamente liberati ed assegnati ad altre compagnie. La Lombardia non può attendere oltre, il Paese non può attendere oltre, perché Malpensa è strategicamente inserita in tutti i corridoi plurimodali. È indispensabile un piano di sviluppo delle infrastrutture di trasporto integrato con gli aeroporti per garantire e velocizzare la mobilità delle merci e delle persone. Il corridoio dei due mari, quello che unisce Rotterdam a Genova attraverso Sempione e Novara, il Corridoio 5 - quello storico - tra Lisbona e Kiev, il corridoio 1 tra Berlino e Palermo: Malpensa è veramente il nodo cerniera in questa cornice. L'Europa finanzia le grandi opere infrastrutturali fino al 20 per cento dei costi di investimento e il CIPE nel 2001 ha approvato una serie di interventi infrastrutturali che insistono su Malpensa: e ora, cosa succede? Succede che Alitalia sceglie Fiumicino, ma lo fa con la lentezza fastidiosa del pachiderma e con la complicità e l'indecisione cronica del Governo. Siamo convinti che il Governo abbia pesanti responsabilità sia nella drammatica situazione in cui versa Alitalia, sia nel tentativo di sopprimere Malpensa, altrimenti non si spiegherebbe l'atteggiamento folle di Palazzo Chigi, che, fino a prova contraria, detiene il 49,9 per cento di Alitalia. Perché avete perso tempo con Airone, anziché tessere rapporti di diverse proporzioni? Quale sarà il deprezzamento di Alitalia sul mercato senza l'*hub* della Malpensa? Perché Alitalia, partecipata dallo Stato, non ha rilanciato proponendo acquisizioni anziché solo dismissioni? Tutto lasciava intendere che, visto il ruolo stabile di Alitalia su Fiumicino, dovesse essere proprio Malpensa a risentire maggiormente della crisi del vettore nazionale. Il Governo non ha pensato allo sviluppo coordinato degli scali italiani secondo ruoli strategici - come dicevo prima - ben definiti, destinando anche le relative risorse. Il Governo ha chiuso entrambi gli occhi per continuare nella tutela irresponsabile degli insostenibili privilegi corporativi di Alitalia e di parte dei suoi dipendenti. Il Governo gioca la partita, il Governo non fa l'arbitro, e non riconosce l'ovvio, cioè quello che di positivo dice il mercato su Malpensa e di negativo su Fiumicino. Gli studi relativi alla crescita del trasporto aereo sostengono che il traffico passeggeri del Nord d'Italia passerà nel giro di sedici anni dai 49 milioni del 2004 a 101 milioni del 2021; oggi Malpensa è il quinto *hub* d'Europa con 38 destinazioni servite; il traffico è cresciuto, tra il 2002 e il 2006, del 23,8 per cento, di cui ben l'11 per cento solo nel 2006, ossia il doppio rispetto alla media europea. Senatore Paolo Brutti, di solito ci differisce solo una consonante, qui invece ci differisce tutto: capisco e ho tutto il rispetto per Perugia, ma Milano non è Perugia e la Lombardia non è l'Umbria; quindi o suoi numeri vanno forse rivisti, certamente favore dell'*hub* di Malpensa. Vogliamo parlare anche del traffico merci? Nessun problema: tra il 2002 e il 2005 è cresciuto del 39 per cento, con nuovi voli cargo per scali strategici per il futuro, come Taipei, Kuala Lampur, Abu Dhabi, che vanno ad aggiungersi agli scali cosiddetti tradizionali. Non so se si è capito, ma Malpensa - lo dico anche con orgoglio - può fare a meno di Alitalia, ma occorre mettere la Regione Lombardia e l'aeroporto stesso nelle condizioni di poter agire rapidamente, affinché Malpensa e l'indotto da esso, generato non abbia contraccolpi negativi. Malpensa chiede efficienza e decisioni per poter resistere autonomamente in un'area geografica che produce il 31 per cento del PIL nazionale e dove è attivo il 24 per cento delle aziende, che generano il 47 per cento dell'*import* e il 41 per cento dell'*export* della nostra intera Nazione. Del resto, la sola Lombardia concentra nei propri confini il 36 per cento di imprese italiane con partecipazione in imprese estere. Stiamo parlando di 900 aziende e di 206.000 addetti. Ma come abbiamo detto, non è però un *derby* tra Roma e Milano. Dobbiamo solo snocciolare dati oggettivi e articolare analisi obiettive per capire la miopia nella scelta di Alitalia e quindi del Governo Prodi, che ne detiene 49,9 Del resto la scelta strategica di ridurre drasticamente Malpensa sembra dettata da ragioni più politiche che industriali ed è per questo che impegniamo il Governo a sbloccare tutte le opere già approvate dal CIPE e collegate direttamente o indirettamente a Malpensa, affinché infrastrutture all'avanguardia possano attirare altre compagnie, oltre che sviluppare economia. Impegniamo il Governo anche sotto il profilo delle relazioni internazionali, affinché vengano rivisti gli accordi extra UE, nella direzione di garantire la designazione e l'operatività multipla di vettori italiani e comunitari e la possibilità per vettori intercontinentali di operare direttamente su Malpensa. Impegniamo il Governo a decidere in fretta sul futuro di Alitalia allettando il mercato internazionale, perché - come abbiamo detto - Alitalia senza un forte radicamento nel Nord del Paese è destinata ad un ruolo marginale. Con una solida *partnership* il vettore potrà svilupparsi, evitare licenziamenti, ingloriosi ridimensionamenti, ma soprattutto garantire lo sviluppo dell'*hub* di Malpensa, con tutto ciò che di positivo ne consegue per l'economia nazionale e il territorio lombardo. la sfida alla competitività dell'intero Paese nel settore dei trasporti e dei collegamenti, piaccia o meno, passa anche e soprattutto dallo sviluppo dell'*hub* intercontinentale di Malpensa. onorevoli colleghi, Malpensa ha incassato lo sfregio politico di questo Governo. Chiede solo di potersi difendere e rilanciare sul mercato europeo e mondiale. Le potenzialità ci sono e il dispositivo delle nostre mozioni mira a salvaguardare da pericoli incombenti, che sono la confusione, l'indecisione e la disorganizzazione che stanno piegando Alitalia ed il sistema aeroportuale italiano. In conclusione, signor Presidente, preannuncio che la dichiarazione di voto a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale la svolgerà il senatore Martinat. Mi sento di poter dire sin d'ora che noi fonderemo le nostre - consentitemi il termine - mozioni di bandiera con quelle della Lega, del senatore Castelli, che è d'accordo; voteremo ovviamente le nostre mozioni di bandiera e successivamente quella sottoscritta dai colleghi della Commissione trasporti.

mi auguro, anche se gli aspetti prodromici della discussione ne hanno già dato un segnale, che questo dibattito non si esaurisca in una sterile contrapposizione tra Nord e Sud

quanto questa visione sarebbe, nel caso fosse insidiata in qualcuno di voi, controproducente e miope per la possibilità, l'entità e l'incidenza di un territorio così ricco di opportunità e di contributo alla composizione del PIL del nostro Paese. Sarebbe miope cercare di penalizzare quel territorio attraverso scelte che giudico chiaramente non percorribili.

Desidero solo riprendere la definizione che di questo piano è stata data dal presidente Prato, cioè un piano di sopravvivenza e di transizione. Mi chiedo, e chiedo a voi, se tale definizione sia compatibile con il ridimensionamento di Malpensa, con la *mission* di sopravvivenza e transizione, o se, invece, questa scelta in realtà non nasconda altri obiettivi. Voglio citare una ricerca, secondo me piuttosto significativa, redatta dallo Studio Ambrosetti, che stima che l'attuazione del piano industriale presentato il 30 agosto dall'Alitalia bloccherebbe nel 2015 il traffico a Malpensa a 26 milioni di passeggeri, con una perdita per l'economia locale stimabile in 15 miliardi di euro, a fronte di una possibile crescita fino a 42 milioni di passeggeri, qualora lo scalo si sviluppasse a pieno regime, che porterebbe alla creazione di circa 15.000 posti di lavoro in più, con un incremento di 25 miliardi di fatturato (visto e considerato che alcuni colleghi facevano valutazioni di tipo aziendalistico nei confronti del tema Alitalia-Malpensa). A fronte di uno scenario di questo genere, è evidente - lo Studio Ambrosetti è uno studio terzo, di conseguenza non tacciabile di essere di parte - per quale motivo, nel presentare un piano di salvataggio, di transizione - diciamo così da parte dell'Alitalia si vuole penalizzare Malpensa. Credo che qualche motivazione, a mio modesto modo di vedere le cose, ci sia e sia per certi versi preoccupante. La mia opinione è che per collocare sul mercato Alitalia,

Nord Italia è molto appetibile. Oltretutto, nel momento in cui si dovessero finalmente realizzare tutte le infrastrutture previste dal piano sottoscritto dai vari Governi, il bacino a due ore da Malpensa si allargherebbe - questo potrebbe succedere entro il 2012 - a circa 17 milioni a circa 17 milioni di passeggeri. In buona sostanza, credo che le compagnie che sono interessate ad acquisire Alitalia abbiano un fortissimo interesse nei confronti di quel bacino, di conseguenza abbiano chiesto ad Alitalia di stralciare l'*hub* del Nord per poterlo acquisire. Compagnie come Air France, come Lufthansa, ma le stesse compagnie della British Airways chiaramente vogliono acquisire Alitalia o sono disposte ad acquisire Alitalia però senza quel bacino, perché quel bacino è di loro interesse commerciale e lo vogliono naturalmente acquisire nel pacchetto complessivo di Alitalia. Di conseguenza, per ottenere questo risultato, il piano di ristrutturazione dell'Alitalia ha sacrificato la cosa secondo loro più semplice e non invece una sana e magari anche difficile ristrutturazione aziendale, che sarebbe la strada da perseguire, nel tentativo di ridurre i costi

pleonastico e finanche inutile sottolineare la gravità della situazione che investe la compagnia di bandiera (io la chiamo ancora così). Siamo di fronte a un disagio che si protrae da tempo e fin troppo avvezzi a considerare Alitalia affetta da una malattia cronica, una sorta di perenne degente, tanto che il piano industriale per il triennio 2008-2010 suona come la campanella che annuncia l'ultimo giro, recitando - com'è noto ampiamente - linee guida che si traducono in misure atte a garantire la sopravvivenza e la transizione. Non v'è alcun dubbio che non possa darsi transizione senza sopravvivenza, ma sarebbe miope in tal caso risolvere tutto in un tirare a campare che condurrebbe sicuramente al baratro. Problemi complessi esigono risposte complesse; anche i tagli alle spese e naturalmente gli eventuali sprechi, se non accompagnati da un progetto di ampio respiro, non costituiscono una risposta reale e duratura. Non dobbiamo dimenticare che al destino di Alitalia è legato il destino di migliaia di lavoratori, dunque di famiglie, e che pertanto soluzioni radicali si ripercuoterebbero in maniera significativa. Ma dobbiamo anche cercare di uscire da una prospettiva di strumentalizzazione politica, e lo dico a qualche collega della maggioranza. A far tempo da un anno, infatti, il futuro di Alitalia e il dualismo tra Malpensa e Fiumicino continuano ad infiammare il dibattito sia politico sia mediatico. L'ottimizzazione delle infrastrutture e dei servizi non si risolve dentro il paradigma di una contrapposizione Roma-Milano, che equivale nei temi e nei toni assunti da taluni in uno scontro Governo-opposizione. Mi corre l'obbligo ricordare, anche se da parte di qualche collega del centro-destra ho sentito in Aula oggi valutazioni

non mi pare che sia stato fatto granché o che siano stati affrontati i nodi che sono poi venuti al pettine. È troppo facile oggi dare la croce addosso solo al Governo, come se il disegno sotteso a detta sopravvivenza e transizione si riducesse ad un incremento e alla valorizzazione di Fiumicino a scapito di Malpensa. Tuttavia, il problema c'è ed è reale; inutile negarlo. Può darsi che alcune valutazioni mosse alla nascita del nuovo *hub*, pensato come infrastruttura eminentemente europea, con particolare riferimento al traffico merci e passeggeri del Sud Europa, si siano rivelate solo parzialmente efficaci. è pur vero che, a fronte dei dati di cui siamo in possesso e malgrado i problemi infrastrutturali, solo in parte risolti (penso, per esempio, alla rete stradale e ferroviaria), Malpensa ha registrato un significativo tasso di crescita in Europa che, salvo errore, risulta essere il più alto in assoluto con il suo 25 Mi domando se non sia un errore smantellare, anche se solo in parte, una intrapresa di questa entità, una struttura che ha comunque inanellato, e sarebbe sciocco negarlo, solo nell'anno solare 2007, una serie importante di risultati e riconoscimenti. Mi domando altresì se non sia opportuno, prima che necessario, favorire una serie di misure che garantiscano una continuità di crescita e l'acquisita competitività di Malpensa nel più ampio quadro del sistema aeroportuale italiano. Potare radicalmente una pianta equivale ad abbatterla; è chiaro che operare in una diversa direzione comporti un prezzo e che sia imprescindibile perseguire un modello aziendale più duttile, al passo con i tempi e con la concorrenza del mercato. L'avvenuta mancanza di una risposta chiara rispetto al primo bando di gara per la cessione del pacchetto azionario pubblico, che si è concluso senza esito, fa riflettere; cercare delle soluzioni interne di investimento e di rilancio. Non suoni come un discorso di parte perché non siamo in presenza di una questione settentrionale che ci si limita ad evocare e sventolare come una clava per denunciare le inadempienze dell'Esecutivo. Obiettivamente, occorre, una volta di più e in senso generale, manifestare anche in questa circostanza attenzione e, soprattutto, maggiore e concreta sensibilità nei confronti della parte trainante, dal punto di vista produttivo ed economico del Paese, non in una logica di sterile e anacronistica rivendicazione strettamente territoriale - oggi qualcuno ha detto campanilistica - ma in una prospettiva razionale che sappia valorizzare intelligentemente aspirazioni ed oggettive potenzialità nell'interesse più ampio di tutta la comunità nazionale. Sulla questione Alitalia le responsabilità sono molte e le domande cui non si è stati in grado di rispondere affondano ormai nel passato; migliorare Malpensa, la sua forza-lavoro e le sue potenzialità, significa valorizzare, non solo un'area nevralgica della piccola, media e grande impresa e dei suoi occupati, ma l'Italia nel suo complesso: una via, dunque, non semplicemente consigliabile, ma necessaria e in qualche misura vincolata.

ho ascoltato con grande attenzione il dibattito fin qui svolto, e credo davvero di poter affermare che il Governo comprende e in larga misura condivide le preoccupazioni espresse in questa Aula circa il futuro del settore del trasporto aereo nel nostro Paese, un settore cruciale per l'economia e le esigenze di mobilità dei cittadini; allo stesso modo però il Governo, anche nella sua veste di azionista di maggioranza relativa, nutre una profonda preoccupazione per il futuro della principale compagnia italiana, Alitalia. Del resto, le valutazioni del Governo sul piano industriale di Alitalia recentemente annunciato non possono prescindere da un'analisi oggettiva e realistica del posizionamento competitivo e finanziario della società, anche alla luce delle problematiche che investono il settore del trasporto aereo e di quello aeroportuale in Italia. Proprio al fine di consentire una valutazione pienamente articolata, non parziale o distorta, dell'orientamento del Governo, consentitemi quindi di ripercorrere quanto accaduto nei mesi scorsi, a partire dalla decisione, assunta nel dicembre del 2006, di cedere il controllo di Alitalia, avendo constatato l'impossibilità di realizzare uno stabile e proficuo risanamento dell'azienda nel contesto attuale, un contesto caratterizzato innanzitutto da anni di risposte inadeguate, da parte non solo dell'azienda ma anche del Governo e delle organizzazioni sindacali, alla crescente concorrenza del mercato, in un contesto di presenza pervasiva della politica; e ancora un sistema aeroportuale estremamente frammentato e, in alcuni casi significativi, penalizzato da infrastrutture di collegamento carenti; e ancora una regolamentazione inefficiente e spesso non trasparente; e, da ultimo, una elevata frammentazione e conflittualità sindacale. Pertanto, la cessione del controllo dell'azienda a soggetti in grado di consentire ad Alitalia di perseguire il necessario rafforzamento industriale, competitivo e finanziario, beneficiando allo stesso tempo di auspicabili sinergie operative, è apparsa la via naturale, nonché probabilmente obbligata, per la salvaguardia della società e degli interessi generali del Paese. Tale scelta - ricordo - è stata generalmente condivisa e, per quanto riguarda il Governo, la determinazione in tal senso viene confermata con convinzione. Quali erano, e sono dunque, gli obiettivi che il Governo intende perseguire attraverso la cessione del controllo di Alitalia? In primo luogo - come ho accennato - quello di affidare la gestione della società a soggetti industriali e finanziari capaci dal punto di vista imprenditoriale e dotati di adeguati mezzi finanziari e patrimoniali, impegnati a realizzare un importante piano industriale di risanamento, sviluppo e rilancio di Alitalia. In secondo luogo, il Governo ha posto al centro della propria iniziativa il perseguimento di ineludibili obiettivi di salvaguardia dei profili di interesse generale: adeguata offerta dei servizi e copertura del territorio; livelli occupazionali coerenti con le iniziative industriali programmate; mantenimento dell'identità nazionale della società, del suo logo e del suo marchio; stabilità del futuro assetto azionario. E' con questi obiettivi, dunque, che il Ministero dell'economia lo scorso dicembre ha avviato la procedura di vendita; una procedura che necessariamente doveva essere impostata e svolgersi nel pieno rispetto della normativa che, in particolare, prevede che la dismissione di partecipazioni dello Stato venga condotta con modalità trasparenti e non discriminatorie. La procedura di vendita, inoltre, non avrebbe potuto prescindere dai vincoli derivanti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato (per cui non è possibile - ad esempio - conferire una cosiddetta "dote" alla società posta in vendita) e dalla necessità di assicurare in ogni caso la piena autonomia gestionale ed imprenditoriale dei soggetti coinvolti, anche se controllati dallo Stato (e penso ad Alitalia stessa, a Fintecna e ad Alitalia Servizi). Non intendo ripercorrere in dettaglio le diverse fasi della procedura, ma solo brevemente soffermarmi a chiarire un aspetto che da molte parti è stato indicato come la principale causa del suo esito negativo. Il Governo avrebbe infatti imposto ai potenziali acquirenti una serie di "paletti", così numerosi e di entità tale da impedire l'emergere di seri e concreti interessi da parte del mercato. Ebbene, in questa sede posso con serenità esprimere la convinzione che, se si analizzano con obiettività i vincoli che il Ministero ha ritenuto di prevedere nell'ambito della precedente procedura, sarà generalmente convenuto che le finalità sottostanti - i cosiddetti requisiti di interesse generale - appaiono allo stesso tempo opportune e legittime. In estrema sintesi, venne richiesto all'acquirente del controllo di Alitalia: innanzitutto un impegno a perseguire quanto lo stesso acquirente avrebbe indicato nel proprio piano, come necessario per il risanamento e il rilancio dell'azienda e, quindi, indirettamente, nel proprio interesse, non quindi un obbligo di effettuare scelte aziendali e operative indicate dal Governo; un impegno ad assicurare la salvaguardia dell'identità nazionale (intesa come mantenimento della sede della società in Italia, del marchio, del logo e del portafoglio dei diritti di traffico); ed ancora un impegno a non cedere la partecipazione acquisita per un periodo di 3 anni; infine, un impegno a mantenere non i livelli occupazionali attuali o quelli minimi che il Ministero avrebbe potuto individuare in via autonoma, ma unicamente i livelli che lo stesso acquirente avrebbe ritenuto congrui in relazione alle iniziative previste nel piano e, quindi, tali da risultare coerenti con gli obiettivi di risanamento e rilancio dell'azienda. Purtroppo, però, l'esito delle procedura è stato - come noto - negativo. Non solo i principali operatori europei del settore hanno ritenuto di non partecipare alla procedura ma soprattutto, tra i soggetti che invece vi hanno preso parte, nessuno ha presentato un'offerta vincolante. Ciò nonostante, il Governo ribadisce la ferma intenzione di realizzare tempestivamente la cessione del controllo di Alitalia, nella convinzione che questo sia l'unico percorso capace di condurre ad un risanamento stabile dell'azienda, sia sotto il profilo competitivo che finanziario. Sulla base di tale convincimento, lo scorso 31 luglio il Ministero dell'economia ha designato il dottor Prato quale nuovo presidente di Alitalia ed ha espresso l'auspicio che il nuovo vertice aziendale «provveda a individuare tempestivamente soggetti industriali e finanziari disponibili ad acquisire il controllo della Società» e ad assumere l'impegno a «promuovere il risanamento, lo sviluppo e il rilancio di Alitalia, tenendo conto dei profili di interesse generale ritenuti imprescindibili da parte del Governo in un'ottica di continuità e adeguatezza di servizio del trasporto aereo in Italia». Il Ministero, infine, si è riservato di valutare «con piena disponibilità le modalità tecniche di cessione del controllo che la Società formulerà ai propri azionisti». Allo stesso tempo, ed anche allo scopo di creare le necessarie condizioni di contesto, il Governo ribadisce la propria disponibilità ad intraprendere le più opportune iniziative per rendere maggiormente appetibile l'operazione, sia con riferimento alla particolare situazione dell'azienda (si pensi in tal senso all'effettiva concessione di ammortizzatori sociali, come annunciato lo scorso mese di maggio), che a quella del settore industriale di riferimento, avviando una politica di sviluppo razionale che riguardi tutte le aree del Paese e tutti i protagonisti del settore, ad iniziare dal sistema aeroportuale. In tale ambito il Governo è impegnato alla tempestiva definizione dell'annunciato piano degli aeroporti ed alla realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano, in primo luogo Malpensa. Nel passare, nello specifico, al piano industriale recentemente approvato dal consiglio di amministrazione di Alitalia, ritengo sia opportuno soffermarmi sulle motivazioni che hanno indotto la società a predisporre un nuovo piano industriale, avendo ritenuto che tale adempimento non fosse ulteriormente procrastinabile. Fino allo scorso mese di giugno, infatti, l'azienda, considerata la procedura di vendita in corso da parte del Ministero dell'economia, non aveva ritenuto di effettuare la revisione del precedente piano industriale e aveva rinviato ogni ulteriore valutazione al riguardo ad una data successiva all'acquisizione di tutti gli elementi necessari. In seguito, preso atto del mancato esito della procedura di vendita da parte del Ministero dell'economia, la società, già prima del rinnovo del vertice aziendale, aveva ritenuto ormai non più procrastinabile l'impostazione di un nuovo documento programmatico, che definisse tempestivamente le più opportune iniziative in grado di contenere l'emorragia patrimoniale e finanziaria che continua a indebolire l'azienda ed inoltre assicurasse l'imprescindibile mantenimento dei presupposti di continuità aziendale, il cui venir meno determinerebbe una rapida accelerazione nella già grave situazione finanziaria di Alitalia. Nella impostazione delle linee guida del nuovo piano industriale, l'azienda, in particolare il nuovo *management*, ha comunque sempre evidenziato come lo stesso si incardini nel più volte confermato intendimento del Governo di cedere il controllo di Alitalia, risultando quindi, come lo ha definito la società, un piano di transizione e sopravvivenza, in attesa che si realizzi l'ingresso del nuovo azionista di controllo. Ma se la definizione di un piano industriale da parte di Alitalia e l'intendimento del Governo di cedere il controllo sono, come detto, strettamente connessi, capire e sottolineare che i ruoli della società e del Ministero azionista sono, e devono essere, ben separati e differenti. Alitalia, infatti, è una società quotata, soggetta a obblighi informativi e di comportamento vigilati dalla CONSOB. Gli amministratori devono operare per il perseguimento degli interessi, non del socio pubblico di riferimento, ma esclusivamente della società e, quindi, di tutti gli azionisti. Sono infatti tenuti, con responsabilità diretta e personale, a rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e a perseguire unicamente finalità economiche. Tornando ai contenuti del piano industriale di Alitalia, rilevo che gli obiettivi di fondo che lo stesso intende perseguire siano senz'altro condivisibili. Tali obiettivi possono così essere riassunti. Innanzitutto, modifica e ridimensionamento dell'assetto di *business* della compagnia nel periodo transitorio, in modo da renderlo più sostenibile da un punto di vista economico, in un contesto di migliore efficienza operativa. Poi, salvaguardia del valore del *brand* Alitalia attraverso la ridefinizione della missione industriale e di un profilo competitivo distintivo. Infine, miglior posizionamento industriale così da favorire l'ingresso di soggetti terzi in possesso di competenze specifiche e risorse finanziarie da destinare allo sviluppo della compagnia. È inoltre confermata l'esigenza di un consistente apporto di risorse finanziarie, mediante aumento di capitale. In tale visione complessiva, quindi, il piano appare del tutto coerente, sia con l'esigenza di definire le più opportune iniziative, da avviare nel più breve tempo possibile, per preservare il valore dell'azienda e rallentare il *trend* di perdite e di erosione della liquidità, sia con il percorso confermato dal Governo per la tempestiva individuazione di soggetti industriali e finanziari disponibili ad acquisire il controllo della società.

in questi termini. Questa situazione, oggettivamente problematica sotto il profilo industriale e competitivo, accompagnata alla gravissima crisi finanziaria della società, ha dunque indotto Alitalia a predisporre un piano industriale di «sopravvivenza e transizione». Naturalmente il piano potrà e dovrà essere oggetto di modifiche e implementazioni in relazione alle scelte di tipo industriale che il nuovo azionista di controllo di Alitalia intenderà effettuare. Del resto, va sottolineato come il piano, ad eccezione di alcune prime e propedeutiche azioni, si avvierà sostanzialmente dalla prossima stagione estiva, ovvero a partire dall'aprile 2008. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, che spero abbiano evidenziato come il piano di Alitalia sia volto prioritariamente a consentire il contenimento delle perdite e quindi ad assicurare la sopravvivenza dell'azienda, nell'attesa che si completi il processo di cessione del controllo, il Governo esprime parere contrario sulla mozione 1-00135, presentata

con la precisazione che il quinto capoverso del dispositivo, così come riformulato, debba essere inteso come un impegno di Alitalia a rendere disponibili gli *slot* non appena non le saranno più necessari..

a condizione che venga espunto il quinto capoverso delle premesse dalle parole: «la situazione...» fino a «...criteri di mercato;» e venga, inoltre, riformulato il quarto capoverso del dispositivo come segue: «a dare applicazione al regolamento europeo CEE 95/93 e successive modificazioni, attivandosi affinché vengano sentite le Regioni per l'assegnazione degli *slot* negli scali ricadenti sul territorio regionale».

Attiro ora l'attenzione dei colleghi sulla decisione che dobbiamo prendere a questo punto: sulla base dei tempi che erano stati predeterminati, dovremmo sfondare di molto il termine di chiusura della seduta, che è fissato alle ore 13,30. In questo caso non saremmo in grado di votare alcuna mozione.

di ridurre drasticamente i tempi di ciascun intervento in sede di dichiarazione di voto. In questo modo potremo concludere attorno alle ore 13,30 le dichiarazioni di voto per passare poi alle successive votazioni, votazioni, in ogni caso, sfondando il termine delle ore 13,30 per la chiusura della seduta, ma in questa seconda eventualità di poco. La Presidenza, quindi, propone una riduzione di tre minuti per ogni dichiarazione di voto, dando facoltà naturalmente ai colleghi che lo intendessero fare,

Signor Presidente, colleghi, gli indirizzi del Governo in materia e il piano industriale dell'azienda recentemente varato impongono di completare il processo di risanamento di Alitalia, predisponendo al tempo stesso un nuovo modello aziendale più efficiente e rigoroso. Questo, in sintesi, il senso della mozione firmata tra gli altri anche dal sottoscritto, nella quale si chiede al Governo di avviare subito una politica organica sul nostro sistema del del trasporto aereo con interventi anche legislativi equilibrati e mirati alla piena valorizzazione delle diverse aree del Paese. Numerose polemiche hanno di recente riguardato le scelte del piano industriale di Alitalia 2008-2010, relative al ridimensionamento dei voli della nostra compagnia della nostra compagnia di bandiera, dallo scalo di Malpensa a favore di Fiumicino. Tali polemiche non sembrano essere suffragate dai fatti, in quanto, per stessa ammissione del consiglio di amministrazione, questo piano industriale dovrebbe essere solo un piano di sopravvivenza, e transizione e la scelta di ridurre i voli intercontinentali a Malpensa è dettata dal fatto che, come ha ammesso anche lo stesso ministro Bianco, la nostra compagnia di bandiera è un vettore che ha deciso di cancellare solo temporaneamente i voli dallo scalo milanese, perché ha problemi a far quadrare il bilancio, tra l'altro, già ampiamente deficitario. Allo stato attuale Allo stato attuale delle cose, per sviluppare Malpensa non si può contare su questa Alitalia, semmai si deve considerare una nuova prospettiva. È quello che chiediamo al Governo di fare, impegnandolo con la mozione sottoscritta, che punta a un non più rinviabile e razionale sviluppo di tutto il sistema aeroportuale italiano nel quale possano trovare pieno sviluppo anche le potenzialità dello scalo di Malpensa. Per questi motivi noi del Gruppo dei Popolari-Udeur, fiduciosi, in quanto auspicato in merito dal Governo, esprimiamo il nostro voto favorevole. il sistema dei trasporti in Italia, sia aereo che ferroviario, ha provocato costi aggiuntivi al bilancio statale ben superiori ai costi della politica, e questo è un dato statistico ben preciso e, ovviamente, senza alcuna valenza giustificativa. Le mozioni al nostro esame non risolvono certamente questo grave problema dei costi del trasporto in Italia. Si tratta a nostro avviso della causa principale, dal quale discendono tutti i problemi ai quali le mozioni danno, in gran parte, risposte accettabili e suffragate del senatore Castelli - da dati statistici oggettivi, che non possono essere assolutamente disattesi da scelte politiche superficiali. Il futuro del trasporto aereo risiede ormai, ed è un dato generalmente condiviso,

Il sistema dei trasporti in Italia è oberato poi da costi aggiuntivi del trasporto, pari ormai a circa un quarto della finanziaria, che questa mattina è stata illustrata, forse con troppa enfasi, in quest'Aula. Le conclusioni sono le Le conclusioni delle mozioni sono in buona parte apprezzabili, soprattutto si agirà decisamente nel senso di lasciare libero il trasporto in Italia di operare secondo logiche del mercato. Il Gruppo La Destra si asterrà quindi sulla mozione Mazzarello, dove abbondano meri auspici sul futuro dello scalo Malpensa, mentre una mozione di maggioranza dovrebbe contenere impegni ben precisi, e voterà a favore di tutte le altre mozioni illustrate in quest'Aula.

allora io alle ore 13,30 tolgo la seduta. La questione è molto semplice. Pensavo fosse interesse, in particolare, non l'ho detto, del Gruppo che lei presiede,

Signor Presidente, è davvero incredibile che le macerie di Alitalia rischino di travolgere una cosa seria, una struttura importante qual è l'aeroporto di Malpensa. Devo dire che sono rimasto deluso anche dalla miopia di alcuni colleghi e dal basso profilo di certe considerazioni che hanno rappresentato esigenze di carattere provincialotto e territoriale dimenticando una cosa fondamentale, che Malpensa non è soltanto un aeroporto lombardo, non è nemmeno solo un aeroporto italiano, ma è una infrastruttura *hub* voluta dall'Unione Europea. Non a caso, quando nel 1994 al Parlamento europeo votammo i 14 progetti prioritari del cosiddetto Gruppo ad alto livello Christophersen, Malpensa era l'unico progetto aeroportuale

era una struttura strategica per il reticolato dei collegamenti aerei europei. Cadono dunque tutte le considerazioni provincialotte legate al *derby* Roma-Milano o Fiumicino-Malpensa, collegate a interessi magari importanti, ma piccoli e nazionali. Non si può distrarre l'attenzione dell'Europa da una realizzazione ormai compiuta. Va detto che ci sono altri colleghi che erano come me al Parlamento europeo in quel momento a sostenere Malpensa e a dibattere sulle argomentazioni e non fu nemmeno molto difficile far passare il progetto di Malpensa per due ragioni. Da un lato, infatti, tale progetto richiedeva uno stanziamento finanziario

(non si può trattare un tema così delicato come fosse un caso isolato), cioè di quello delle grandi linee transeuropee. Quando nel 2003, sotto la Presidenza italiana, queste grandi linee furono ampliate ottenemmo anche altre tre realizzazioni che ci riguardano: il Corridoio dei due mari Rotterdam-Sempione-Novara-Genova, il Corridoio 5 Lisbona-Torino-Milano-Trieste-Kiev ed il Corridoio 1 che parte da Berlino, passa da Monaco, da Verona e arriva fino a Palermo. Ebbene, anche questi corridoi furono immaginati e progettati in maniera strategica pensando a Malpensa come collegamento. Casomai, adesso occorre completare questo piano di collegamenti infrastrutturali con quelle opere che il CIPE nel 2001 ha indicato come funzionali al potenziamento di Malpensa, vale a dire l'accessibilità generale dell'*hinterland* milanese, la Torino-Milano-Verona-Venezia, l'asse ferroviario Milano-Genova, l'asse stradale pedemontano lombardo e l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano. Quindi, non solo non è assolutamente accettabile che con il pretesto del disastro Alitalia si riduca l'importanza di Malpensa come aeroporto strategico europeo che guarda ben oltre il profilo delle Alpi e i *derby* nazionali, ma occorre accelerare la realizzazione di queste opere. Quanto poi alla fruibilità,

non è vero. Nel mio piccolo, i miei 200 voli l'anno, negli ultimi trent'anni, li ho fatti. Bisogna capire ciò che si afferma e non ragionare partendo soltanto dalla provincia. Quanto alla funzionalità perché non c'è confronto. Se proprio vogliamo scendere in campo per quanto riguarda i voli intercontinentali, Malpensa vince 18.000 contro 5.000 nei confronti di Fiumicino: il 76 contro il 24 per cento. Evitiamo questi confronti fratricidi. In Italia - lo ha detto ancora una volta l'Europa - possono coesistere due grandi aeroporti *hub*, quello di Malpensa e quello di Fiumicino, ma a patto che ripeto - i disastri interni di una società di bandiera come l'Alitalia non travolgano Malpensa. Per quanto riguarda il risanamento di Alitalia, molti colleghi autorevoli hanno espresso diverse proposte. Mi unisco a una su tutte: quella di rivedere il numero sicuramente esagerato di dipendenti. Non c'è il tempo e non è questo il luogo per fare un'analisi tecnica ma, partendo dalla nostra piccola esperienza quotidiana, un ammaestramento lo possiamo portare a casa. Tutti noi facciamo settimanalmente la spola su Roma, venendo dai nostri collegi e dalle nostre residenze. Cominciamo a guardare i voli interni, che non superano quasi mai un'ora di tragitto, a volte 40-50 minuti. Ebbene, vi sono sei persone che, durante il viaggio, ci offrono un bicchiere d'acqua oppure un caffè. *(Applausi dal Gruppo* *LNP).* È veramente indispensabile avere a bordo di questi aerei interni sei persone? Non riusciamo a resistere un'ora senza un caffè? Credo proprio di sì. Due persone basterebbero per aiutare i passeggeri a sistemare il bagaglio, mentre le altre potrebbero essere opportunamente impiegate in altre mansioni. Cominciamo da queste piccole cose e potremmo immaginare davvero una razionalizzazione complessiva globale, ma non con le indicazioni date dal nuovo amministratore delegato, che ha partorito tante idee, ma nessuna con coraggio. ci vuole coraggio e determinazione, in primo luogo per sanare una situazione e poi per pensare al riordino di tutto il resto del sistema. Ma non si tocchino le cose che funzionano, e Malpensa è tra queste.

delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli e quelli delle Province di Trento e Bolzano si sono incontrati, evidenziando l'emergenza infrastrutturale del Nord. Hanno chiaramente posto l'emergenza sul sistema aeroportuale, indicando Malpensa come *hub* principale e fondante di tutto il sistema. Penso che da qui bisogna ripartire, con grossi investimenti su Malpensa, proprio dal punto di vista infrastrutturale. Bisogna che Malpensa sia raggiungibile in modo umano da Bologna, Venezia, Torino, da altre parti d'Italia e dal Nord Europa, perché possa davvero assolvere al proprio compito, sul quale abbiamo investito tanto denaro e su cui abbiamo patito tanti costi ambientali. Il tema dello sviluppo di Malpensa quindi mi pare sia centrale. In questo caso penso che sia molto ben evidenziato il tema dalla mozione n. 144, sulla quale noi del Gruppo Per le Autonomie esprimiamo voto assolutamente favorevole. Rispetto al tema di Alitalia, penso che sia utile andare verso uno svincolo del piano industriale di Alitalia da Malpensa, proprio per garantire a tale aeroporto la possibilità del pieno sviluppo delle sue potenzialità industriali.

ma necessarie. Condividiamo l'iniziativa del Governo Prodi per evitare il fallimento dell'azienda con la ricerca di un alleato industriale e finanziario, mettendo sul mercato le quote azionarie pubbliche. Tale compito è affidato al nuovo presidente dell'azienda che ha presentato il nuovo piano industriale, piano che indiscutibilmente ridimensiona i voli su Malpensa e taglia alcuni voli intercontinentali. Si tratta di un difficile piano di tagli, ma indispensabile per evitare il rapido fallimento dell'azienda Alitalia.

perché riconosce che bisogna separare il destino di Malpensa dal destino di Alitalia, altrimenti affonderanno insieme. È evidente che l'aeroporto di Malpensa, collocato in un'area economica, industriale, insediativa, strategica e di alta valenza del nostro Paese, ha una forte capacità di attrarre e produrre traffico di queste settimane di molti operatori privati del trasporto aereo che si sono candidati a sostituire i tagli di Alitalia lo dimostra - anche come scalo di valenza internazionale e questa separazione tra il destino di Alitalia e il destino di Malpensa consentirà a Malpensa il proprio autonomo sviluppo in un'area europea ormai di mercato del trasporto aereo liberalizzato. Voglio ricordare ai colleghi, soprattutto a quelli della maggioranza, che sarebbe un obbligo normativo, se Alitalia non utilizzasse più gli *slot* che oggi detiene ed esercita, la messa sul mercato di queste tracce orarie evidentemente, ma sarà indispensabile comunque inquadrare Malpensa in una strategia integrata dei trasporti nel bacino padano, migliorare le infrastrutture, in particolare - aggiungo da ambientalista - quelle ferroviarie, di accesso e regolare il complesso degli aeroporti che offrono servizi ai cittadini e alle imprese in un'area importantissima del del nostro Paese. Andrà inoltre applicata, come chiede la mozione, una valutazione ambientale strategica, che, ricordo, è ormai un obbligo normativo da anni, a seguito dell'applicazione di una direttiva europea relativa agli interventi sugli aeroporti, quindi non solo su Malpensa ma sull'intero complesso degli aeroporti, finalizzata anche alla riduzione dell'inquinamento e dell'impatto ambientale; da stime recenti, il trasporto aereo emetterebbe circa il 10 per cento delle emissioni di CO2 a livello mondiale, ma il traffico aereo è completamente detassato e non paga alla collettività i danni che genera, nemmeno in minima parte. Anche il traffico aereo quindi ha dei limiti e ha dei limiti anche di espansione; e anche di questo dobbiamo tener conto nel confronto sul futuro del trasporto aereo e di Alitalia nel nostro Paese. Nella mozione c'è anche - lo voglio sottolineare - un richiamo importante al recupero di relazioni industriali e criteri di gestione del personale che sappiano motivare i lavoratori, che dovranno responsabilmente essere attori di questo difficile piano industriale, un piano che si rende indispensabile per il salvataggio dell'azienda, ma richiede anche responsabilità e concertazione con i lavoratori, che saranno quelli direttamente toccati da questo nuovo piano industriale. quindi concludere annunciando il voto favorevole del Gruppo dei Verdi alla mozione Mazzarello ed il voto contrario alla mozione presentata dalla Lega, perché riteniamo non colga il vero problema del futuro di Malpensa, innanzitutto, e richiamando ad un forte equilibrio tutti noi per evitare inutili e sbagliate contrapposizioni tra Roma e Milano ma per l'adozione di una strategia equilibrata, ambientalmente sostenibile, economicamente efficiente del trasporto aereo nel nostro Paese.

vorrei insistere, nonostante quello che hanno detto alcuni colleghi, su questo fatto: sei passeggeri su dieci, con origine e destinazione Milano, usano aeroporti alternativi a Malpensa e caricano gli *hub* di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Madrid nell'ordine. Nove passeggeri su dieci, con origine e destinazione il Nord Italia, si servono di aeroporti alternativi a Malpensa: anche qui gli *hub* Francoforte, Parigi, Madrid, Roma, Monaco e Amsterdam. Al di là di tutto quello che si dice, tecnicamente Malpensa non è oggi ancora diventato un *hub* nel senso vero della parola. In altri termini, i vettori europei dicono ai milanesi e ai viaggiatori dal Nord Italia: fatevi trovare a Malpensa o a a Malpensa o a Verona a quell'ora che vi porteremo a Francoforte, Amsterdam, Londra, da dove andrete nel resto del mondo. Questa è la situazione reale; se non si affronta questo problema, Malpensa è destinato - più rapidamente per via della crisi Alitalia, meno rapidamente se si risolve la crisi Alitalia - ad entrare in una situazione ingovernabile.

e ci sono pochi vettori intercontinentali diretti che li portano via, non si può seguire - è la mia opinione - una via dirigista, che avrebbe un impatto quantitativo importante solo riducendo drasticamente i cosiddetti voli punto punto dalle altre città del Nord Italia - 86 destinazioni nazionali, 251 destinazioni internazionali dal resto degli aeroporti dell'Italia del Nord - ed eliminando drasticamente i vettori *low cost*, che sono cresciuti negli ultimi cinque anni in Italia del 48 per cento, mentre i *full service carrier* - tra i quali rientra Alitalia - sono cresciuti solo del 2,4 Ora è in campo una proposta della Ryanair per l'utilizzo di Malpensa: è interessante, ma i grandi vettori non scalano in una base di armamento totalmente in mano a compagnie *low cost*, bisogna saperla questa cosa prima di caldeggiare una soluzione di questo genere. Bisogna fare una scelta strategica impegnativa, che nessuno può compiere al posto del gestore aeroportuale di Malpensa, l'imprenditore industriale che non sa rinunciare, con il comportamento che tiene in questo momento, ad una posizione di rendita. Forse loro pensano quello che è stato detto qui: siamo al centro dell'area più ricca dell'Europa, che porterà in volo 100 milioni di passeggeri; il punto è che questi 100 milioni di passeggeri saltano completamente Malpensa. Quanto al ruolo del Governo, Quanto al ruolo del Governo, credo debba svilupparsi attraverso gli accordi bilaterali di traffico, che però - lo ricordo a chi ne parla con una certa leggerezza - non riguardano i vettori comunitari: i vettori comunitari non sono assoggettati a questi accordi bilaterali di traffico. Gli accordi disciplinano la capacità di traffico, il volume delle frequenze, le compagnie interessate, le condizioni di offerta (quindi anche le tariffe) e, in particolare, gli aeroporti di decollo e di atterraggio. Sarebbe necessaria una diversa regolazione degli *slot*, cioè delle bande orarie di decollo e di atterraggio. In ogni caso, il Governo occorre che operi sul coordinatore dell'allocazione delle bande (capisco che una questione difficile da esprimere), cioè quello che decide gli *slot*, per superare il principio di autorizzazione basato sulla priorità storica a favore di quello dell'utilizzo continuativo: se Alitalia non utilizza più alcuni *slot*, li deve abbandonare al di là del fatto che storicamente sono i suoi. L'assetto dei diritti di traffico ad operare su Malpensa è competenza del Ministro dei trasporti: lo fa attraverso l'ENAC e addirittura su indirizzo del Ministro degli affari Bisogna che questa catena di comando funzioni, si possono bilanciare i pesi di Malpensa rinegoziando e ampliando questi diritti, ma soprattutto verso i vettori non comunitari. Poiché Malpensa, anche se sembra strano, è un aeroporto tecnicamente congestionato, è soggetto alla coordinazione di Assoclearance, che assegna gli *slot* liberi od inutilizzati ai nuovi entranti secondo una percentuale che può essere molto spostata a loro favore rispetto all'attuale percentuale del 50 Questo riporterebbe nell'aeroporto di Malpensa un bene patrimoniale - quello degli *slot* - con cui acquisire nuovo traffico aereo: migliorando il trasporto, rendendo più efficienti i servizi a terra, proteggendo i bagagli e diminuendo le tariffe e le tasse aeroportuali, affidando alle compagnie di gestione alcuni *termin**al*, Malpensa ha tutte le carte in regola per affermarsi come un grande *open airport*, un modello nuovo per tutta l'Europa. E non chiamiamolo «cielo duro», come è stato proposto per le compagnie aeree che lì fanno scalo: chiamiamolo ancora il grande aeroporto di Malpensa.

che mandi in giro per lavoro i propri dipendenti a spese dei dipendenti, quindi non venite a dire che i 400 equipaggi al giorno che vanno in giro lo fanno a spese loro, pagando i biglietti, perché in questo modo prendete in giro il Paese ed anche i vostri elettori. E questo è un altro discorso.

della vendita del prodotto. Dico questo visto che si parlava di aziende, di aeroporti che devono produrre e tutte le altre balle che sono state raccontate. Nonostante questo e che nel piano industriale di qualche anno fa

Questo non lo dico perché sono della Lega o per via del dualismo Milano‑Roma, che non esiste (tanto noi siamo noi e gli altri sono gli altri: non è questo il problema che ci preoccupa), ma nell'interesse di Alitalia. Adesso vi ritirate a Fiumicino, perché avete un piano di sopravvivenza. Benissimo, andrete avanti due anni; fra due anni cosa farete? Quando avrete perso anche il mercato padano, quando Malpensa sarà stata riempita da tutti gli altri vettori seri d'Europa e continuerà a vendere il 70 per cento dei biglietti del mercato nazionale, Alitalia cosa farà nel suo porticciolo di Fiumicino? Si troverà una grandissima struttura, con un quarto del traffico di oggi. Il libero mercato (visto che come Cosa rossa, Unione o PD non ho ben capito come la pensate) è l'unica cosa che non potete governare. Potete farlo per qualche mese, per qualche anno, ma alla fine il libero mercato va da sé. Se i biglietti si vendono a Malpensa, a Milano, in Padania continueranno a vendersi lì: se ci sarà Alitalia, la gente volerà Alitalia, altrimenti volerà con qualunque altra cosa. E state tranquilli che, una volta che Malpensa sarà stata lasciata libera da Alitalia, nel contingente potrà essere un piccolo problema per noi (ed un grande problema ideologico, perché non si sottoscrivono i contratti e poi unilateralmente ci si tira indietro: l'impegno a Malpensa, infatti, è stato sottoscritto), quindi è evidente che oggi Malpensa si troverà con un po' di difficoltà, se di colpo andrà via Alitalia, ma sarà una difficoltà temporanea: tutti quelli che oggi prendono l'aereo per andare a Zurigo o a Francoforte, perché non ci sono i servizi Alitalia a Malpensa, quando troveranno gli aerei che Alitalia a Malpensa non ha mai messo, cominceranno a volare su Malpensa e da 20 milioni arriveremo ai 40‑50 di cui si è detto

Fiumicino quanto costa alla collettività dal momento che viene tenuto in piedi con affitti fasulli di Alitalia che vengono mantenuti dal pubblico erario? Per concludere, ricordiamoci che in Padania c'è l'economia del Paese. Dico queste cose non con supponenza o arroganza, ma per far capire al resto del Paese che, se il modello adottato su scala nazionale è il nostro, il Paese si salva. Diversamente, se continuate a pensare di poter mantenere in piedi un Paese con cittadini di serie A e cittadini di serie B,

avete preteso di mettere sul mercato una compagnia che non ha più aerei, che non ha più un mercato e che ha il triplo dei dipendenti, con la pretesa che chi l'avesse eventualmente comprata

colleghi, la faccenda di Alitalia è molto aggrovigliata. Ne veniamo fuori se abbiamo un principio direttivo chiaro. Il principio direttivo chiaro è che su Alitalia occorrono soluzioni di mercato perché, a termini di legislazione europea, non siamo in grado di fare iniezioni di denaro pubblico a questa il prestito dell'azionista, l'ultima possibilità che abbiamo avuto di sostenere Alitalia; poi ho chiamato i sindacati e le autorità regionali della Lombardia e del e del Lazio e ho detto: guardate che Alitalia andrà in fallimento perché siete tutti convinti che non potrà fallire e che lo Stato interverrà, ma lo Stato non potrà più intervenire; ci vogliono soluzioni di mercato. Capisco che gli amici della Lega non sono molto convinti che questo piano industriale contenga soluzioni di mercato; e devo dire che condivido i loro sospetti. Tuttavia, "soluzioni di mercato" significa che non è il Parlamento che giudica il piano industriale. Il piano industriale è una direzione aziendale che si assume la responsabilità di dargli esecuzione ed è meglio un cattivo piano industriale che nessun piano industriale. Per tanti anni, infatti, la dirigenza di Alitalia ha avuto il vincolo di non mollare Malpensa, di non mollare Fiumicino, di non fare la società per i servizi a terra

mercato vuol dire mercato per tutti. Ora, c'è il sospetto che si voglia tagliare le ali a Malpensa per favorire l'ulteriore decollo di Alitalia. Questo non è consentito, non è possibile, non è ammissibile e questo Senato non lo può accettare. Senatore Brutti, Malpensa è il quinto *hub* d'Europa: quello che lei dice è vero, in parte. Noi abbiamo fatto due *hub* e contemporaneamente abbiamo varato una legislazione che non ha fatto sistema con gli altri aeroporti, puntando sul punto a punto anziché sull'*hub.* Se desidera recarsi a Strasburgo deve passare da Parigi. In Italia lei può andare in qualunque parte del mondo partendo dall'aeroporto più piccolo. Non abbiamo fatto una legislazione di sistema ed è una colpa che inizia con il Governo Prodi, non quello di adesso, quello di prima. Però attualmente la situazione è così e Malpensa sta riuscendo egualmente a qualificarsi come un grande *hub* europeo senza compagnia di bandiera che regga il grosso del peso dell'*hub.* Dobbiamo aiutarlo.

Dobbiamo impegnare il Governo nazionale a sostenere l'infrastrutturazione compiuta di Malpensa, che si trova all'incrocio dell'asse Nord-Sud ed Est-Ovest, che sono i due assi fondamentali di infrastrutturazione europea.

la quale era chiaramente destinata al fallimento perché formulata in condizioni non di mercato. Nessuna azienda che avesse buon senso e che non contasse su patti politici sotterranei poteva prendere Alitalia a quelle condizioni. Mantengo la valutazione politica,

abbiamo previsto «coinvolgendo le Regioni nell'assegnazione degli *slot* e delle bande orarie modificando la normativa vigente che assegna questo compito esclusivamente ad Assoclearance». Ci viene proposta un'altra formulazione, sostanzialmente equivalente, che io accetto; accettandola però, ribadisco alcuni aspetti. Il Governo ha paura di parlare di Assoclearance; invece è evidente che, se coinvolgiamo le Regioni e diamo attuazione al regolamento, dobbiamo rivedere una normativa che dà una esclusiva ad Assoclearance. Vorrei dire al senatore Brutti che il nostro problema non è di chiedere ad Assoclearance di essere buona e di rivedere le bande; noi dobbiamo andare verso un sistema nel quale gli *slot* vengano assegnati a chi porta più traffico nell'aeroporto.

che contiene ciò che forse è stato tolto in virtù della richiesta del Governo: non è ammissibile che ci siano comportamenti anticoncorrenziali e taglino le ali a Malpensa; il mercato deve valere per tutti. il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ha già ampiamente espresso la sua posizione sulla problematica generale relativa alla situazione dell'Alitalia. Abbiamo già detto che il trasporto aereo negli ultimi anni è stato interessato da cambiamenti incessanti in direzione della forte liberalizzazione e da una progressiva deregolamentazione che desta in primo luogo preoccupazione in ordine alle ricadute sulle condizioni dei lavoratori e sulla sicurezza e la qualità dei servizi ai passeggeri. Solleva, a nostro giudizio, forti dubbi rispetto agli effettivi vantaggi che ci sembrano in generale tutti da dimostrare. Riteniamo comunque che il risanamento di Alitalia debba essere volto debba essere volto a mantenere un ruolo autonomo di Alitalia nell'interesse del Paese, e in questo contesto non possiamo cavalcare la contrapposizione tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino. A nostro avviso, l'aeroporto di Malpensa deve essere inserito in una logica di sistema rispetto agli altri scali aeroportuali del Nord, anche attraverso il completamento degli interventi infrastrutturali necessari, ma non certo con ulteriori espansioni e potenziamenti che preoccupano i comitati dei cittadini e delle associazioni che vivono su quel territorio. Auspichiamo che il Governo non rinunci a svolgere un ruolo di programmazione per un razionale sviluppo di tutto il sistema aeroportuale italiano, definendo il piano degli aeroporti all'interno del quadro generale del Piano dei trasporti, e garantendo comunque la valutazione ambientale strategica relativa agli interventi sugli aeroporti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento e all'attenzione sull'impatto del territorio, come tra l'altro è specificato nella mozione del centro-sinistra. Auspichiamo altresì che il Governo metta in campo tutti gli strumenti perché si tenga conto delle esigenze dei lavoratori in termini di tutela dei livelli occupazionali, di qualità del lavoro e di superamento della precarietà. Poiché molti di questi contenuti sono stati

credo che i problemi siano essenzialmente due. Uno si chiama Alitalia, e il primo vero nodo di Alitalia è di essere una compagnia area con pochi aerei e troppi dipendenti. È questo il primo dato fondamentale. Il secondo dato, che riguarda invece Malpensa, è essenzialmente uno, Presidente, perché non si può predicare bene e razzolare male: Malpensa nasce come *hub* del Nord - non ripeto quello che è stato detto da altri dei passeggeri, e così via - ma nasce anche come cattedrale nel deserto. Il Governo Berlusconi aveva introdotto tre grandi linee di comunicazione: la Genova‑Rotterdam, la

il Governo Prodi cancella le tre concessionarie che devono costruire il sistema Alta Velocità Genova-Novara-Milano e Milano-Verona-Padova; il tribunale di Genova condanna il Governo a ripristinare le concessionarie e invia il tutto alla Corte di giustizia europea perché ripristini quel ripeto - è il primo dato. Allora, se Malpensa è stata costruita come una cattedrale nel deserto, e con il Governo Berlusconi si stavano attivando i collegamenti, è evidente che, nel momento in cui questo Governo cancella quei collegamenti e non dà la possibilità ai piemontesi, ai veneti, agli emiliani e ai lombardi stessi, di raggiungere l'aeroporto di Malpensa, esso ha difficoltà a decollare. Tutto ciò premesso, credo che uno dei dati fondamentali sia l'accordo che non è mai stato fatto, ma più volte sollecitato, tra Alitalia e Ferrovie dello Stato.

Questo è uno dei nodi: le Ferrovie dello Stato cosa fanno? Forse per la cattiva gestione delle Ferrovie stesse, non si costruiscono le tratte ad Alta Velocità; quando le si costruirà, bisognerà studiare questo sistema. Alcuni casi già ci sono; la Torino-Novara già funziona,

della Torino-Zurigo, della Torino-Parigi, della Torino-Francoforte, perché mi è più comodo, in quanto per arrivare a Malpensa occorrono due ore con la macchina. Ma se ci fosse un servizio di questo genere, credo che i piemontesi utilizzerebbero molto volentieri Malpensa.

Commissione, ha affermato di voler rendere immediatamente disponibili gli *slot* non più strettamente necessari al traffico di Alitalia, senza utilizzare il periodo di sospensione di norma accordato. Spero che ciò avvenga.

quindi, il servizio ai cittadini non si rende, ma si difende la compagnia di bandiera. Noi siamo contrari a questo sistema. Siamo in un libero mercato, e se gli *slot* che l'Alitalia metterà in immediata libertà a Malpensa verranno presi da compagnie *low cost* o da altre compagnie di bandiera, ben venga. Non è questo il problema. Il problema è che bisogna essere competitivi. Tornando alla battuta iniziale: più flotta e meno dipendenti, mentre oggi abbiamo più dipendenti e meno flotta. L'Alitalia deve diventare una compagnia vera, e non semplicemente un rifugio di dipendenti che sono stati «accasati» spesso per motivi clientelari. Del collega Mantica ho apprezzato - come altri del nostro Gruppo

prendo la parola cambiando però il mio primario intervento, che era basato su aspetti tecnici, e quindi mi scuserò se conterrà qualche aspetto polemico. polemico. Oggi abbiamo assistito - ahimè - ad una Italia divisa in due. Altro che federalismo! Siamo ancora all'Italia delle camarille. Siamo ancora all'Italia dove si fanno discorsi estremamente provinciali, dove il mercato non viene considerato, dove ognuno può dire qualsiasi cosa. Si può sfondare con dei dati che sono totalmente falsi o quantomeno non meditati. Ho sentito dire qui che il problema dell'Alitalia è Malpensa e quindi bisogna provvedere a fermare, a tarpare le ali a Malpensa per non far fallire Alitalia. Voglio ricordare - studio i bilanci di Alitalia da qualche anno - che Alitalia è fallita da qualche anno. È fallita per suoi bilanci che hanno avuto una ricapitalizzazione - ahimè falsa, nel senso che è stata una sovvenzione per una inefficienza, una incapacità di gestione, e quindi anche una sovrastima di dipendenti che non sono in Alitalia stessa ma in tutte le società satelliti, non sono altro che società con dei protettorati politici di sinistra, e devono tenere in piedi un sistema che non è più accettabile in un Paese moderno. È chiaro che il sistema del trasporto costituisce un asse fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese. È chiaro anche che nei prossimi vent'anni il traffico aereo sarà raddoppiato. È chiaro che il collo di bottiglia di due *hub* è un aspetto estremamente importante, proprio per la configurazione del nostro Paese, Paese, che è molto lungo e ha due aspetti fondamentali: la capitale e la politica a Roma, ma ma i dati che vi darò adesso (e in ogni caso già ricordati da alcuni miei colleghi) spezzano il Paese in due, nel senso che la vera produttività e la creazione del prodotto interno lordo è al Nord. Quindi, non è possibile pensare che Malpensa debba essere messa in un angolino e che i cittadini del Nord possono venire a Roma. Non verranno mai a Roma a prendere

un aeroporto congestionato. Perché che cos'è Fiumicino? Fiumicino è un aeroporto - e noi tutti lo frequentiamo - con ritardi medi da 30 a 60 minuti. Ha gli aerei sempre in linea. Ha una sporcizia incredibile. È un aeroporto assolutamente mediorientale Quindi, non possiamo accettare questa possibilità. L'attuale bacino di riferimento di Malpensa

Ricordo che Malpensa ha il massimo record di incremento per il trasporto delle merci. Con questi dati non è possibile liquidare Malpensa con delle battute del tipo «il cielo duro». Perché, il «penitalia» è bello? Non capisco per quale motivo nell'Aula del Senato si debba arrivare a simili basse contestazioni, non tenendo in considerazione che il Nord è il fattore trainante di questo Paese... con tutto il rispetto, con tutta la dignità e con tutta la fratellanza, di un federalismo che se non va avanti dimostra ancora la nostra assoluta provincialità e incapacità, tendendo solo a sprofondare verso il Mediterraneo del Sud. È vero anche che l'efficienza operativa ed un sistema di trasporto nazionale sono le due leve per la competizione delle nostre merci.

Noi ci auguriamo quindi, perché abbiamo capito che ormai questa *lobby* è talmente forte, che arrivi qualche compagnia asiatica o degli Emirati arabi. Dico questo perché Air France ha il suo *hub*, e Francoforte ha il suo hub.

che il nostro sistema paese, abbia la forza, la voglia e, soprattutto, la saggezza di considerare che si possono avere due

mandare avanti con grande energia il risanamento e la ristrutturazione di Alitalia, e allo stesso tempo lavorare con intensità, con forza risolvendo i problemi, perché Malpensa resti e diventi un grande *hub* intercontinentale.

su Malpensa come grande *hub* intercontinentale, fondandone le ragioni su una compagnia, Alitalia, che è in crisi fortissima Mi sembra proprio un errore di impostazione dell'Alitalia. Sinceramente credo che finalmente si sia imboccata la strada giusta, non più quella che abbiamo seguito fin qui.

nel ruolo, nella forza della compagnia, che ha continuato a perdere e che ha ridimensionato sempre di più il suo ruolo sul mercato.

Finalmente ci si vuole mettere mano, con una linea nuova, con un indirizzo nuovo, quello che il Governo ha impostato e che il piano industriale

Malpensa è stata un'intuizione importante, grande: quella di avere una *hub* nella zona più ricca del nostro Paese, in una delle aree più importanti d'Europa, dove ci sono le aziende che commerciano, dove vi sono gli scambi anche dal punto di vista del ruolo che Malpensa ha per le merci. Dobbiamo lavorare per confermare tale ruolo, per rafforzarlo, ma non ci possiamo nascondere di fronte alle difficoltà se non vogliamo solamente fare propaganda. Non possiamo arrabbiarci se qualcuno ci dice che i passeggeri, provenienti da Milano, che volano su voli intercontinentali, per il 60 per cento

Ma non è responsabilità della ristrutturazione di Alitalia. È chiaro? Se non vogliamo fare solamente propaganda, dobbiamo porci questi problemi: i problemi delle infrastrutture e degli *slot*. Abbiamo insistito anche

uno schieramento più largo di quello della maggioranza o, comunque, al di fuori delle contrapposizioni maggioranza e opposizione. Per questa ragione, voteremo no alla mozione Castelli, sì alla mozione Buttiglione e sì al dispositivo della mozione Cicolani.

saranno messe ai voti secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'esito di ciascuna votazione non sarà ostativo alla votazione degli strumenti successivi, che si intenderanno messi ai voti per le parti palesemente non precluse né assorbite.

Noi non abbiamo affatto voluto votare interamente la parte del dispositivo che impegna il Governo, perché non siamo d'accordo.

votare le premesse separate dal dispositivo. Presidente, mi scusi, ma visto questo fraintendimento (noi infatti abbiamo tutti inteso in questo modo e non capisco come ciò sia potuto accadere), vorrei correggere il mio voto come voto contrario e vorrei che tutti facessero una dichiarazione contraria perché c'è stato un fraintendimento. Vorrei che fosse messo a verbale che il mio voto è contrario alla mozione n.

interpretate in maniera diversa, però reputo anche politicamente importante che si dia atto in quest'Aula che il voto favorevole espresso dal Gruppo Forza Italia (poiché sono tra quelli che hanno segnalato di votare favorevolmente) riguardava esclusivamente il primo capoverso e che quindi gli altri ci trovano contrari, perché non siamo d'accordo sul loro contenuto sostanziale. È bene che ciò si sappia, perché sappiamo bene che la comunicazione esterna può valere come un consenso del nostro Gruppo o di altri a un'indicazione che invece non condividiamo. Senatore Pastore, non ci sono dubbi, dopo gli interventi della senatrice Alberti Casellati e il suo intervento, sul parere contrario del Gruppo di Forza Italia alla seconda parte della mozione n. 144 (testo 2), di cui è primo firmatario il senatore Mazzarello. Pregherei però i colleghi, quelli che dirigono i Gruppi e tutti gli altri, di seguire con maggiore attenzione i lavori d'Aula

mi rimetto alle sue valutazioni e alle sue decisioni. L'unica cosa che mi permetto di sottolineare è che abbiamo assistito a tante votazioni un po' anomale,

Matteoli, sono talmente d'accordo con lei che, come ho detto prima dell'inizio della votazione, mi sono permesso di annunciare alle colleghe e ai colleghi, quindi anche a lei, autorevole presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, che su questo modo di procedere tutti dovremmo riflettere, proprio per rendere più trasparente e tranquillo il nostro

vedano il proprio voto cambiato in negativo. Se lei non lo fa, credo abbia un atteggiamento assolutamente arbitrario, perché non è logico che io abbia chiesto una votazione difforme e separata per votare allo stesso modo: è la logica qui che soccorre, non l'interpretazione. Non è suscettibile d'interpretazione alcuna; quindi, trovo arbitrario che lei mi abbia tolto la parola e abbia adottato un'interpretazione non plausibile. Chiedo che lei mi risponda nel senso che il voto di Forza Italia venga cambiato secondo quella che era l'intenzione vera di Forza Italia. Senatrice Alberti Casellati, non mi costringa per la seconda volta a toglierle la parola, lei sta sindacando decisioni del Senato della Repubblica, cosa che non ha diritto di fare in alcun modo a norma del nostro Regolamento, per cui le tolgo la parola. Procediamo dunque alla votazione della mozione n.

Burlando. Finché la vicenda è calda e ha un significato e anche forse per chiarire il comportamento del presidente della giunta regionale Burlando, ne solleciterei l'iscrizione all'ordine visto che ci sono anche interpellanze al riguardo di altri colleghi, il più presto possibile; se possibile, nella seduta di interrogazioni della prossima settimana.

*(FI)*. Signor Presidente, so benissimo che qui bisognerebbe urlare, ma anche se parlo a bassa voce è per dire

Pare a me, che ho vissuto prima nella Germania federale, come corrispondente della RAI, il problema della *Rote Armee Fraktion* e i delitti che ne conseguirono quello delle contro le Brigate rosse, quando anche da quella parte venivano definite «sedicenti Brigate rosse», o uomini manovrati da Fanfani per far vincere i *referendum*... Onorevole Presidente, pregherei almeno di avere la sua attenzione. L'indignazione L'indignazione è forte, sentita e motivata per ciò che è avvenuto in questi giorni, con la concessione di benefìci premiali ad un terrorista che non si è pentito; del resto, persone che non si sono pentite o che per lo meno vantano ancora la loro appartenenza ideologica e culturale alle azioni delle Brigate rosse le troviamo in Italia come cattivi maestri che continuano a parlare e a scrivere. Credo soltanto in Adriano Sofri, devo dirlo molto francamente,

e ha mantenuto in carcere fino all'ultimo giorno coloro che si erano resi responsabili di orrendi delitti. Credo che anche noi, proprio sul piano europeo (visto che dobbiamo attuare un coordinamento generale, soprattutto nella lotta contro il terrorismo internazionale), dovremo opportunamente modificare almeno una parte della giurisdizione premiale, quando questa

che ho depositato esattamente due mesi fa, ma che per ragioni formali è stata pubblicata l'11 settembre scorso, dunque quasi un mese fa. Con essa segnalavo il fatto,

che parla tanto di sicurezza in questi giorni, se lo ritenga un fatto normale e, altrimenti, di sapere chi abbia la responsabilità di aver consentito un fatto simile. Un fatto particolarmente preoccupante, leggendo che in questi giorni, in Afghanistan, sono stati

Ho l'onore di essere stato minacciato di morte in aula dal Piancone solo perché mi era stato conferito l'incarico di difenderlo d'ufficio. Quando chiesi il decreto di citazione, questo signore mi disse «Le tirerò due pallottole nella testa», quello che non ha potuto fare ieri, perché gli si è inceppata la pistola.

ha ritenuto che il recupero morale e civile del reo possa verificarsi e che non ci siano limiti alla possibilità della redenzione di chiunque abbia commesso qualunque reato.

che deriva dalle modalità con le quali si è comportato; non formalmente in carcere per avere benefici, perché è questione puramente burocratica e personalistica, ma se il magistrato, nell'esaminare le questioni, abbia visto qual è il grado di pericolosità sociale di una persona. Molte volte invece - lo dico anche per esperienza professionale alla richiesta segue soltanto una valutazione puramente formale. Ora, siamo qui in Senato, l'Aula è mezza vuota e mi spiace di disturbarla proprio ora. Lei sa che uso con una certa parsimonia il diritto di parola, poichè mi piace di più ascoltare che parlare, tanto è quasi inutile molte volte; pertanto, desidero dirle con tutta sincerità che il problema deve essere affrontato in termini di realismo. Il principio deve essere sacro perché è costituzionalmente protetto, il realismo accede al principio con un criterio contemporaneo di moderazione e di considerazione, che molte volte, poichè poichè la Repubblica italiana è basata sul lavoro ma anche sui timbri, consente ad un magistrato di salvarsi l'anima e liberare i corpi di quelli che possono ancora fare del male alla società. Pensiamoci tutti insieme prima di andare a mangiare.

Non mi associo, signor Presidente, al coro di quanti vogliono in questo caso crocifiggere la magistratura, perché sembra un po' come sparare sulla Croce rossa: spariamo sulla magistratura addebitandole la responsabilità di quello che è accaduto, come se la magistratura fosse effettivamente responsabile. Voglio ricordare che i tribunali di sorveglianza in Italia emettono ogni anno innumerevoli pronunce in cui concedono la semilibertà ai detenuti: non fanno notizia queste concessioni, ma fa notizia il caso Piancone. Credo che il problema non vada limitato il problema sta - come si diceva una volta - a monte: è più responsabile il magistrato che concede un beneficio a chi ne ha formalmente diritto, o è più responsabile il Parlamento che ha messo quel magistrato in condizione di emettere quel provvedimento?

a ragione - che si carichino i giudici di responsabilità e poi che li si crocifigga; ai magistrati che, in applicazione delle norme, riconoscono benefìci ai detenuti si richiede - caro senatore Biondi - una difficile prognosi sulla condotta che questi terranno. Non è giusto - e lo condivido - attaccare un giudice sulla base di ciò che è successivamente accaduto. Il problema - cerchiamo di intenderci - non è difendere o attaccare i magistrati, ma cambiare - anche se lei non è d'accordo - la legge Gozzini. Cambiamo la legge Gozzini. Presenti, il Governo, un disegno di legge per modificare quelle norme che consentono ai magistrati di adottare quei provvedimenti e ai Piancone di turno di commettere reati.

dove sono stati annullati una serie di concorsi, poi rimessi a bando, e dove con atto proprio il direttore generale di quella stessa Azienda, prima di andarsene, si è aumentato lo stipendio. Quindi, chiedevo se rientrava nelle disposizioni di controllo sulla spesa finanziaria e sul rientro della Regione Lazio. Siccome in questa finanziaria è previsto un nuovo contributo straordinario per le Regioni che versano in una grave situazione finanziaria, mi sembra eccessivo che i direttori generali, prima di andare in pensione, provvedano ad aumentarsi lo stipendio.

dai colleghi Selva, Biondi e Berselli, relative alla vicenda dell'ex terrorista Piancone, mi permetto - data anche la delicatezza della materia - di suggerire ai colleghi, magari attraverso un'iniziativa tipica del sindacato ispettivo, di

sono in discussione anche il rispetto delle norme vigenti, a cominciare dalla legge Gozzini, alla quale ha fatto giustamente riferimento poco fa il collega Berselli. Senza sindacare nella maniera più assoluta le iniziative della magistratura, si tratta ovviamente, con un atteggiamento molto pragmatico, di valutare concretamente le circostanze e i modi attraverso i quali certe certe vicende si possono verificare. Quindi è materia da investigare e da analizzare. Sarà importante una valutazione, qualora riuscissimo a farla nei tempi più brevi qui in Senato.